per tutte le votazioni da effettuare nel corso della seduta. Onorevoli senatori, com'è tristemente noto, si è spenta la senatrice Lidia Brisca Menapace, da alcuni giorni ricoverata per Covid nell'ospedale della sua Bolzano. Donna brillante, intelligente, forte e di grande determinazione. La sua vita è stata il racconto emozionante di tante battaglie vissute da protagonista, in nome di quegli ideali di libertà, giustizia, pace, uguaglianza e pari opportunità che sono i pilastri della nostra democrazia. Giovane staffetta partigiana, durante gli anni drammatici della Resistenza non volle mai toccare un'arma, ma questo non le impedì di conquistare conquistare il grado di sottotenente e il brevetto di combattente per il coraggio dimostrato in più occasioni nel soccorrere e nel salvare vite. Quello stesso coraggio l'ha sempre accompagnata tanto nelle grandi battaglie politiche quanto nell'impegno quotidiano al servizio dei cittadini, specie di chi è più fragile e bisognoso di aiuto. Prima donna a entrare nel Consiglio e nella Giunta della Provincia di Bolzano, fondatrice e firma autorevole del quotidiano «il manifesto», Lidia Menapace è stata per molti anni una delle voci più importanti del femminismo italiano e un simbolo di libertà per tante donne. Instancabile la sua opera per una società veramente di pari opportunità e di pari dignità tra donne e uomini, specie sul fronte dell'accesso all'istruzione e al mondo del lavoro. Le sue armi erano quelle della pazienza, della persuasione e del dialogo. Eletta al Senato nella XV legislatura, Lidia Menapace ha saputo interpretare il mandato parlamentare con grande entusiasmo e passione, dando prova, in ogni occasione, di competenza, rigore e costante apertura al confronto, sempre costruttivo. Una ricchezza di valori che ha contraddistinto anche la sua azione fuori dalle Aule del Parlamento, nella società civile, come testimone e promotrice di una preziosa cultura della pace universale da contrapporre a ogni forma di paura, di violenza e di prevaricazione. Con Lidia Brisca Menapace ci lascia una grande donna, un esempio di umanità, di coerenza e di instancabile fedeltà ai valori della Costituzione, per tutti noi e per molte generazioni. In ricordo della senatrice Lidia Brisca Menapace invito pertanto l'Assemblea a osservare un minuto di silenzio.

L'ordine del giorno reca: «Comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri in vista del Consiglio europeo

Gentile Presidente, gentili senatrici e gentili senatori, il Consiglio europeo del 10 e dell'11 dicembre presenta un'agenda densa densa di temi di elevata priorità per l'Unione europea sia per quanto riguarda la sua coesione, prosperità e stabilità sia per quanto attiene al suo ruolo di attore globale. Il tema centrale rimane la lotta alla pandemia da Covid, su cui è fondamentale che da parte europea provenga un segnale chiaro di coesione. Al riguardo, il Consiglio europeo è orientato a dare impulso politico al mutuo riconoscimento dei test e a un efficace coordinamento europeo sui vaccini, con particolare riguardo alla loro distribuzione. Solo una risposta internazionale ed europea, del resto, può consentire di superare la pandemia, obiettivo a cui l'Italia lavora intensamente, anche nella prospettiva del Global health summit, che ospiteremo il 21 maggio 2021, nel quadro della Presidenza italiana del G20. A tal fine, stiamo lavorando in stretto contatto con la Commissione europea. La dimensione sanitaria della risposta europea al Covid dev'essere costantemente accompagnata da quella economica e sociale. Rimane urgente, a tale scopo, una soluzione che, dando attuazione all'accordo raggiunto in seno al Consiglio europeo del 21 luglio scorso, superi il veto ungherese e polacco e consenta il tempestivo avvio di Next generation EU e del nuovo Quadro finanziario pluriennale. Porrò con la massima determinazione e urgenza l'esigenza che l'ambizioso programma di investimenti e riforme, finanziato con debito comune, per il quale l'Italia si è spesa fin dall'inizio della crisi pandemica, possa essere avviato nel più breve tempo possibile. I cittadini dei ventisette Stati membri non perdonerebbero un segnale che contraddica lo storico accordo raggiunto sull'adozione di strumenti centrali per la ripresa sociale ed economica e che rappresentano un profondo aggiungo, irreversibile - cambiamento di paradigma nelle politiche economiche perseguite dall'Unione europea. Per la prima volta, infatti, questa si è fatta promotrice di politiche espansive, finanziate da strumenti di debito autenticamente europeo e orientate al raggiungimento di strategie condivise e obiettivi comuni. Questa è una risposta evidentemente e radicalmente diversa rispetto a quella posta in essere in passato, quando, di fronte ad altre crisi (pensiamo a quella del 2011), si adottarono scelte ancora fondate su una logica di austerità, ispirate al prioritario criterio del contenimento del debito. Quelle scelte - è la storia che ce lo dice - si sono rivelate inadeguate a ricondurre i Paesi europei all'interno di una prospettiva di autentica ripresa e sviluppo. Aggiungo anche che si sono rivelate tutto sommato inadeguate anche per quanto riguarda l'obiettivo del contenimento del debito stesso. Continuiamo dunque a sostenere gli sforzi della Presidenza tedesca di turno del Consiglio dell'Unione europea e della Presidente della Commissione europea, rivolti a una soluzione rapida di questa situazione di stallo, causata - come ho già ricordato - dal veto posto da Ungheria e Polonia. Vi anticipo peraltro - lo faccio doverosamente, ma con la massima cautela - che, proprio in queste ultimissime ore, sembrerebbe intravedersi uno spiraglio positivo in questo negoziato.

condivisa dai medesimi Paesi interessati, per quanto riguarda la condizionalità dello Stato di diritto. Ovviamente, non possiamo assolutamente rinunciare a quanto già riconosciuto e affermato sul tema, però si tratterebbe di una dichiarazione interpretativa assolutamente compatibile con gli obiettivi e i principi già affermati. Stiamo a vedere, però, lo ribadisco: nelle prossime ore ci sarà sicuramente un'evoluzione in questo senso. Il vertice euro del prossimo 11 dicembre discuterà in particolare il pacchetto di riforme approvato dall'Eurogruppo lo scorso 30 novembre, che consta di tre elementi:

il cosiddetto *common backstop*, e l'accordo sulla valutazione della riduzione dei rischi nell'Unione bancaria. Com'è noto, la riforma del MES, approdata sul tavolo dell'Eurosummit nel nel dicembre 2019, incorporava l'introduzione del *backstop* comune al Fondo di risoluzione unico, a partire però dal 2024. Il Governo italiano ha agito per ottenere l'introduzione anticipata di tale meccanismo, nel presupposto di rispettare alcuni obiettivi di riduzione del rischio bancario. È stato importante procedere in questa direzione, il Fondo di risoluzione unico e il meccanismo di *backstop*, che è a suo sostegno, rappresentano una forma essenziale di condivisione dei rischi al livello dell'unione economica e monetaria, obiettivo cardine per il nostro Paese. era previsto che si procedesse in sequenza: prima la riforma del MES, poi la valutazione dei rischi, infine l'introduzione anticipata del *common* *backstop*, attraverso la riforma dell'accordo intergovernativo, che regola il trasferimento e la messa in comune dei contributi del MES al Fondo di risoluzione unico. Grazie sempre al contributo italiano, l'Eurogruppo ha raggiunto un'intesa, che consentirà di procedere in parallelo: sarà ora compito dell'Eurosummit sancire questo accordo. Procedere fin da subito in via contestuale consente, tra le altre cose, di anticipare l'introduzione del *backstop* all'inizio del 2022,

dello stato di salute del sistema bancario europeo e di quello italiano, che, prima della pandemia, aveva registrato un miglioramento consistente dei propri bilanci. Su tale base è stato possibile raggiungere più facilmente l'obiettivo di un'entrata in vigore anticipata del *backstop*. Resta ovviamente nella piena disponibilità delle Camere, attraverso la procedura parlamentare di ratifica, la scelta definitiva sull'adesione dell'Italia al nuovo Trattato MES, anche alla luce del più generale stato di avanzamento del pacchetto di riforme dell'Unione economica e monetaria.

Se però proviamo ad alzare lo sguardo, volgendo gli occhi verso una prospettiva più ampia, possiamo convenire che per cambiare l'Europa, soprattutto alla luce della drammatica crisi vissuta in questi mesi, sia decisivo ben altro percorso. In quest'ultima prospettiva, valuto che debbano essere riconsiderate, in modo radicale, struttura e funzioni del MES, affinché sia trasformato in uno strumento completamente diverso.

quindi preannunciare che l'Italia, nell'ambito della Conferenza sul futuro dell'Unione europea, si farà promotrice di una proposta innovatrice, che porti a superare la sua natura di accordo intergovernativo, legato a un paradigma che ritengo ormai obsoleto

che certamente offrono maggiori garanzie di trasparenza e democraticità. Il modello al quale ispirarsi, nel costruire a livello europeo gli strumenti di politica economica del futuro, ce

L'accordo di luglio, che apre la strada a un programma di finanziamento di dimensioni straordinarie, che sarà alimentato con le emissioni di debito comune, è un risultato che fino a pochi mesi fa sembrava a molti irraggiungibile, ma che è stato raggiunto grazie a uno sforzo comune, lungo un percorso non privo di passaggi critici. Abbiamo raggiunto questo risultato muovendoci sempre con spirito costruttivo e affidandoci alla forza degli argomenti e delle proposte. Quest'accordo, insieme al sostegno senza precedenti fornito dalla Banca centrale europea, attraverso il programma straordinario di acquisto di titoli pubblici e privati, sta cambiando oggettivamente la fisionomia dell'intera Unione europea Governo, siamo determinati a lavorare affinché la nuova Europa superi definitivamente l'approccio angusto dell'austerità e abbracci la strada dello sviluppo sostenibile, dell'inclusione sociale, della transizione energetica e dell'innovazione digitale per un'economia europea ancora più competitiva, ma anche più equa, con particolare riguardo, ad esempio, al versante dell'armonizzazione fiscale. Il Governo e - ne sono certo - il Parlamento continueranno a lavorare in questa direzione, consci delle difficoltà, ma anche consapevoli dei significativi vantaggi per gli Stati e per gli stessi cittadini europei che possono derivare da un'Unione più salda e più solidale.

Anche Sure, infatti, si fonda sull'emissione di titoli di debito comune europeo a favore di tutti gli Stati membri. Si tratta di progressi che rafforzano l'unità e la solidarietà europea a sostegno della ripresa economica e di una maggiore resilienza dal dal punto di vista economico e sociale. Venendo agli altri temi che sono in agenda per il prossimo Consiglio europeo, fra le priorità connesse alla ripresa economica europea vi è indubbiamente quel *green deal* europeo al quale la Commissione lavora già dalla fase precedente alla pandemia e che impone un consenso pieno sul livello di ambizione dell'Unione in materia di cambiamento climatico e sulle modalità per realizzarlo. è una priorità che l'Italia intende perseguire anche nella prospettiva della conferenza COP26. Sapete che l'anno prossimo avremo la responsabilità, insieme alla Gran Bretagna, di questo che è il più importante evento in materia di ambiente e di clima. È per noi essenziale che quest'obiettivo sia accompagnato dal riconoscimento anche finanziario degli sforzi già sostenuti in questi anni da alcuni Paesi, tra cui l'Italia, per avanzare verso i *target* climatici,

in particolare con l'obiettivo di intensificare, tanto più a seguito dei recenti attentati occorsi in Francia e in Austria, la cooperazione intraeuropea nella prevenzione e nel contrasto al terrorismo. L'Italia è naturalmente concorde e impegnata al riguardo e condivide l'obiettivo di una migliore collaborazione in ambito europeo tra autorità di polizia e agenzie di *intelligence.* Il nostro Paese concorda inoltre con l'azione continentale di prevenzione e di contrasto alla radicalizzazione, anche attraverso la rimozione dei contenuti terroristici in Rete. vostra attenzione - il nesso politico che qualcuno vuole stabilire tra Schengen e immigrazione, che è stato riproposto anche nel dibattito europeo proprio in materia di sicurezza. Quanto alle relazioni esterne, il Consiglio europeo esaminerà diverse questioni di grande importanza, a partire da quella turca. Sulla scorta delle conclusioni del Consiglio europeo straordinario che si è tenuto agli inizi di ottobre e del Consiglio ordinario del 15 e 16 ottobre, anche tenendo conto degli sviluppi degli ultimi due mesi, saremo chiamati a valutare i rapporti con Ankara e le prospettive future.

I segnali verso Ankara dovranno essere chiari, ma non innescare dinamiche di *escalation.* Occorre infatti mantenere una finestra di opportunità per favorire un'agenda positiva, giacché alimentare tensioni non è nell'interesse europeo, a maggior ragione perché stiamo parlando di un Paese che comunque è membro della NATO. Sempre in tema di relazioni esterne, le conclusioni del Consiglio europeo prenderanno atto di una discussione sui rapporti transatlantici nella prospettiva di imprimere slancio, con l'avvento dell'Amministrazione Biden, alla collaborazione tra Unione europea e Stati Uniti. Se infatti riteniamo che gli Stati Uniti, almeno nei primi passi della nuova amministrazione, rimarranno concentrati su priorità interne - penso alla lotta alla pandemia e alla ripresa economica siamo anche convinti che il presidente eletto Biden, come peraltro mi ha confermato nel corso della nostra prima conversazione telefonica, avrà un approccio molto positivo al multilateralismo e ai rapporti transatlantici e sono certo che considererà l'Europa come un *asset* per gli stessi Stati Uniti. Starà comunque all'Unione europea proporre e alimentare un indirizzo politico e un'agenda di lavoro che possano intercettare le priorità americane, in particolar modo con riguardo alle sfide globali della pandemia, del cambiamento climatico e della ripresa sociale ed economica nel segno dell'equità, dell'inclusività e della sostenibilità, peraltro assi portanti del programma della Presidenza italiana del G20, che, come sapete, è appena iniziata. Ancora, tra gli altri temi che sicuramente rientrano tra le priorità americane di comune interesse con l'Unione europea vi è il rilancio del commercio internazionale anche come strumento di crescita, in particolare attraverso la riforma, ormai davvero necessaria, dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) e l'auspicato superamento di dispute e dazi; e ancora, la sicurezza e la difesa, anche al fine di superare finalmente le crisi regionali. Dovremo pertanto dimostrarci determinati a rafforzare il contributo europeo alla sicurezza e allo sviluppo internazionali, in linea con le giuste ambizioni dell'Unione a svolgere un ruolo più forte e visibile nel mondo, ma anche essere chiari e trasparenti con Washington su cosa intendiamo noi europei - che qui dovremo interrogarci con molta attenzione - per "autonomia strategica" dell'Unione europea: dobbiamo declinare questo concetto e caricarlo di significati politici positivi

L'Italia è attivamente impegnata nel rilancio di un partenariato rafforzato e consapevole, fondato su un approccio strategico e un programma concreto di iniziative, come recentemente condiviso al vertice italo-spagnolo il 25 novembre scorso.

Al Consiglio europeo è inoltre prevista la consueta informativa della cancelliera Merkel e del presidente francese Macron sullo stato di attuazione degli accordi di Minsk. L'informativa risponde all'esigenza - che l'Italia ha fatto sempre valere di avere anche una discussione politica fra *leader*, prima di procedere al rinnovo semestrale delle sanzioni economiche settoriali nei confronti della Federazione Russa. Per quanto riguarda

chiedendo sempre di acquisire un aggiornamento sullo stato dell'attuazione degli accordi di Minsk. Vogliamo evitare automatismi: rientra nella nostra capacità di dialogo cogliere e attribuire a qualsiasi sistema sanzionatorio la natura strumentale, evitando che sia fine a se stesso. Ai temi all'esame di questo Consiglio europeo si potrebbe aggiungere anche quello della relazione futura tra Unione europea e Regno Unito a seguito degli ultimi sviluppi negoziali tra Bruxelles e Londra, la cui perdurante distanza su alcuni temi cruciali

punto. Vedremo quale prospettiva concreta si viene a delineare nelle prossime ore. Il nostro quadro di priorità è però molto chiaro. Su questo l'Unione europea si è mossa sin qui in modo encomiabile con una voce sola e con chiarezza anche di indirizzo politico. Tra i temi ancora in discussione abbiamo anche una gerarchia di importanza. Al primo posto c'è senz'altro la necessità di raggiungere un *level playing field*. Noi non possiamo permettere che alcuna forma di partenariato, oggi e domani, possa consentire a un Paese terzo di avvantaggiarsi delle opportunità e delle potenzialità offerte dal mercato comune senza soggiacere alle medesime regole che tutti gli Stati membri rispettano. Questa è la prima priorità. poi un problema di *governance*: dobbiamo fare in modo che eventuali dispute siano risolte in modo chiaro, con un meccanismo certo di risoluzione anche dei conflitti. Infine - sto non a caso indicando un ordine gerarchico di priorità - c'è il tema della pesca, che per molti Paesi è importante. Per noi lo è evidentemente molto meno, ma diciamo che è un tema di rilevante rilievo economico. Una relazione profonda e ambiziosa tra Unione europea e Regno Unito era e rimane nell'interesse di tutti, ma - come sempre abbiamo detto - non a ogni costo. Tale relazione deve essere equilibrata affinché tutte le imprese italiane ed europee possano competere con quelle britanniche in maniera leale. Serve quindi anche una *governance* coerente, che impedisca il ripetersi di situazioni come quelle legate all'*internal market bill* sulla questione nordirlandese. L'Italia, quindi, riafferma il sostegno al capo negoziatore europeo Michel Barnier e al presidente von der Leyen e resta convinta che l'unità tra Stati membri rimanga un passaggio obbligato per tutelare al meglio gli interessi di cittadini e imprese. osservo che, nel quadro di incertezza confermatosi in quest'ultima fase negoziale, risulta ancora più essenziale il lavoro che l'Italia negli ultimi mesi ha intensificato con tutti gli Stati membri e con la Commissione europea per misure di comunicazione e preparazione alla fine del periodo transitorio, così da essere pronti per ogni scenario. Mi avvio a conclusione. La prossima riunione del Consiglio europeo sarà un altro tassello del percorso che stiamo costruendo per affrontare le sfide che attendono il nostro Paese e la comunità di Stati che si è raccolta storicamente sotto l'emblema Unione europea. Sono sfide - voi stessi potete misurarle - molto complesse,

ciascuno per il proprio ruolo e compito, in modo da restituire il senso e la sintesi a un impegno collettivo. Spesso in Aula - lo ricorderete - ho rivolto un appello al dialogo e all'unità alle forze di opposizione in alcuni passaggi devo riconoscere che esso ha trovato ascolto. Rimane sempre quel che ho ribadito in altre sedi e circostanze: il tavolo del confronto con le opposizioni resta sempre aperto, ma è importante anche che ci sia la massima coesione delle forze di maggioranza. È importante parlarsi, così come lo sono il confronto dialettico e la varietà di posizioni, la varietà di posizioni, nonché superare, in una sintesi superiore, con spirito costruttivo, la varietà di opinioni, perché non dobbiamo mai disperdere le energie. Dobbiamo sempre concentrarci sugli obiettivi che ci stanno a cuore e che giustificano la nostra presenza qui e la nostra azione. La coesione delle forze di maggioranza ci consente - stiamo parlando di un prossimo Consiglio europeo e di un futuro importante per l'Europa - di continuare a battersi in Europa. Vi assicuro che ci metterò tutta la più ferma determinazione nel fornire il giusto contributo critico e anche il coraggio necessario a sostenere un programma di riforme come quello in corso e anche il processo di rinnovamento che si preannuncia per le istituzioni europee. Tra un po', infatti, inizierà la Conferenza sul futuro dell'Europa, nella quale dovremo misurare la nostra capacità di incidenza, la nostra energia rinnovatrice

Signor Presidente, senatrici, senatori, Governo, oggi siamo chiamati a esprimerci su più di una modifica: la riforma del Meccanismo europeo di stabilità e la ratifica dell'Accordo intergovernativo sull'attivazione del *common* *backstop*. È stato impossibile reperire il testo ufficiale della riforma. Inoltre, dal documento a disposizione in Aula compare un ordine del giorno in cui la riforma del MES occuperebbe una posizione tra le varie ed eventuali. I punti all'ordine del giorno del Consiglio europeo sono: Covid-19, cambiamenti climatici, sicurezza e relazioni esterne. Mi chiedo come mai oggi non ci si trovi in quest'Aula a riflettere su temi come la situazione del Mediterraneo orientale o la Turchia. Ma veniamo a noi. Ciò che ci viene chiesto di avallare o meno con un unico voto richiederebbe, in verità, l'espressione della volontà senatoriale in due distinte operazioni. La riforma del MES incorpora l'introduzione del *common backstop* al Fondo di risoluzione unico, prevista a partire dal 2024, anticipandola al 2022. Tale anticipazione prevede che sia effettuata preventivamente una valutazione sulla riduzione del rischio bancario. Concordo con le valutazioni positive operate dalla BCE e dal Comitato di risoluzione unico in merito alla situazione delle esposizioni deteriorate - i famosi *non-performing loan* (NPL) - e alla capacità di assorbimento delle perdite. I risultati vanno verso un'unione bancaria che vede l'Italia già in una posizione avanzata rispetto agli altri Paesi europei in merito all'organizzazione del sistema bancario sulla base di quanto indicato dai trattati europei relativi. Altra questione è la "riforma-non riforma", nella quale si prevede un ingresso facilitato al finanziamento tramite la presentazione di una lettera di intenti, anziché la firma di un *memorandum.*

La conclusione è che il riferimento al *recovery fund* sostanzialmente ha una visione prospettica di di sviluppo futuro, mentre il MES è già superato. Il Parlamento è sovrano; la *task force* si trova già qui. Ci sono dei progetti già pronti e il Parlamento è pronto e chiaramente disponibile a una leale collaborazione.

Al netto dell'emergenza pandemica Covid-19, il tema del MES è stato il più dibattuto in Italia nel corso

caso, presidente Conte, due elementi hanno reso questo dibattito davvero sgradevole. Il primo è quello di cui abbiamo sentito parlare nelle scorse ore, e cioè che il MES fa schifo e noi non lo attiveremo. che cosa sia questo: forse un senso di responsabilità? Secondo me no: questo è un menefreghismo, un opportunismo che ha l'odore acre di poltrone vecchie, di poltrone di Ministeri, di Ministri e anche di Sottosegretari. Il secondo punto è che lei nelle prossime ore parlerà alla comunità europea. Allora mi chiedo, le chiedo e vi chiedo, di quale comunità stiamo parlando, se questa comunità prevede degli strumenti che affondano e affossano i nostri colleghi, fratelli e amici europei.

Dalle vostre parole sembra quasi che l'Europa sia una specie di osteria, una grande osteria che prepara piatti nauseabondi, che tanto noi non ordineremo mai. Siamo preoccupati di questo, del fatto che un nostro collega e fratello europeo tra qualche tempo, tra qualche mese, sarà costretto a ordinare quel piatto nauseabondo e a darlo in pasto ai propri cittadini e ai propri figli.

Abbiamo scoperto che esistono dei veti che non sono più veti. Abbiamo scoperto che esistono dei mandati a Ministri che poi non sono mandati così ufficiali. Abbiamo scoperto che esiste un MES che sta al di sopra di ogni giurisdizione. Allora mi chiedo: forse sono saltate completamente le regole democratiche in Europa e in Italia? Chiudo questo mio brevissimo intervento dicendo semplicemente quello che ho sostanzialmente detto un anno fa. Diremo no al MES, perché vogliamo dire no a quella austerità che non fa rima con comunità. Faccio un appello a tutti i miei colleghi senatori,

ex miei colleghi, che oggi sono in maggioranza, e a tutti quelli che il 5 luglio 2015 volarono in Grecia per sostenere il no della Grecia alla *troika*. Faccio un appello a tutti i miei ex colleghi e a tutti i colleghi, dicendo che quello che conta non è il punto di caduta: quello che conta è l'atterraggio e noi abbiamo paura che voi ci stiate portando a sfracellarci a terra insieme a voi. Quel 5 luglio in piazza Syntagma ad Atene c'erano due *big* 5 Stelle: uno è al di fuori delle istituzioni e si tiene stretto il suo secondo mandato, mentre l'altro ha presieduto stamattina la Camera l'altro ha presieduto stamattina la Camera dei deputati, anche con i voti del centrodestra. Questi due *big* in piazza Syntagma ad Atene dissero:

Signor Presidente, signor Presidente del Consiglio, Ministri e colleghi, anche chi guarda distrattamente i titoli di stampa sa perfettamente che gli ultimi giorni sono stati

sono stati giorni tumultuosi per arrivare a questo dibattito e alla risoluzione di maggioranza,

- ripeto - è piuttosto reticente. E in questa verbosità ognuno leggerà quello che vuole. Questo è il rischio. Alcuni amici dei 5 Stelle leggeranno che comunque intanto è sì, però poi ci vediamo in Parlamento per la ratifica. Questa è un'ovvietà. Non c'è bisogno di scrivere che i trattati poi devono passare in Parlamento, a meno che appunto ci sia il retro pensiero, e cioè che, quando arriverà la ratifica, Altri ci leggeranno una riserva meno perentoria e meno definitiva. Ma vorrei metterla in guardia sul fatto che tutti gli sforzi italiani che lei ha proposto, e che mi sento anche di condividere, non hanno tempi così brevi. Quindi c'è da parte sua un impegno a provarci, ma non può esserci un impegno a non procedere se non c'è la riforma complessiva, perché questo ci porterebbe non dico alle calende greche, ma esattamente così. Il ministro Gualtieri e anche lei sapete perfettamente quanto sarà difficile riformare

di +Europa-Azione abbiamo presentato una risoluzione - che l'avete approvata alla Camera e ve ne ringraziamo - molto più breve, più netta, più chiara. Noi non vogliamo dirle, signor Presidente del Consiglio dei ministri, dei ni. Noi vogliamo dirle dei sì chiari, netti, precisi, senza girarci troppo intorno. Sono convinta che l'Unione europea abbia dimostrato sulla pandemia di essere lungimirante e generosa più di quanto sia stata descritta negli anni scorsi. Se ricordo bene, solo un anno fa bisognava non approvare il MES; adesso sì, ma dipende. Io credo che la forza contrattuale - e voi lo sapete benissimo - stia nell'arrivare con delle posizioni più nette,

alla vigilia di un importante vertice europeo, che riguarda non solo il MES - ci ricordava lei, signor Presidente del Consiglio - ma anche i cambiamenti climatici, l'esito della Brexit, la sicurezza dopo gli attentati terroristici in Francia e in Austria, i rapporti transatlantici dopo le elezioni di Biden. La discussione politica italiana, invece, si è concentrata soprattutto sulla riforma del Meccanismo europeo di stabilità.

per le forze politiche, sia quelle di maggioranza, nostre alleate, sia quelle di opposizione, che hanno approfondito e cercato di capire. Francamente, però, a volte questo dibattito mi è parso sovrattono rispetto al merito.

sono sui tavoli del dibattito dell'Eurogruppo dal 2017. È nella riunione del 13 giugno 2019 che emerge un ampio consenso dell'Eurogruppo sulla proposta di revisione del trattato.

Poteva e può l'Italia, con il ruolo che riveste in Europa, con la scelta europeista che è il tratto fondamentale su cui nasce il Governo che oggi guida questo Paese, Paese, votare contro un accordo che vede tutti gli altri Paesi d'accordo, dopo aver lavorato e contribuito in modo importante a modificarlo in linea con gli interessi italiani?

su cui poi si esprimerà il Parlamento? Alcuni vedono potenziali rischi, io ci vedo delle potenzialità positive. Ma sarà una discussione che faremo nel momento in cui decideremo eventualmente di attivarlo; oggi questa discussione non c'entra con l'ordine del giorno. Francamente credo che molti nostri alleati europei abbiano assistito un po' increduli alla nostra discussione, così accesa e partecipata. e partecipata. Mi auguro che tutti quanti sentano la responsabilità di far capire che l'Italia è un Paese stabile, europeista e che nell'Europa crede. Voi sapete,

la maggior parte di questi progetti sono trasversali. Si è aperto un dibattito surreale e si dice che i Ministeri non contano più niente. Ma sono progetti trasversali che riguardano non solo diversi Ministeri, ma talvolta anche amministrazioni locali. locali. Francamente, che non si preveda che possa essere utilizzato uno strumento come la struttura di missione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri non lo comprendo, mi onoro di aver fatto parte di un Governo presieduto dal presidente Renzi e poi anche di quello di Gentiloni Silveri, e strutture di missione ce n'erano:

che i Ministeri siano coinvolti e che il Consiglio dei ministri sia protagonista. Nessun progetto può andare avanti se si pensa di escludere i Ministeri. È in corso una discussione veramente surreale per chi ha avuto qualche esperienza di Governo,

l'Italia è la Nazione che ne beneficia maggiormente, francamente la preoccupazione di tutti noi dovrebbe essere quella di come predisporre i progetti. So che questa è la discussione che avete fatto in Consiglio dei ministri, e questa è la discussione che dobbiamo fare in Parlamento, perché l'Italia, oggi, di questo ha bisogno.

per il contributo che avete dato in questo periodo all'identificazione e all'affermazione di soluzioni a livello europeo e per i risultati che avete ottenuto nella politica europea sui due fronti che caratterizzano la politica europea di un Paese come l'Italia: quello esterno dei negoziati in sede comunitaria e quello interno, qui in Parlamento e nel Paese. Riferendomi al lavoro fatto in Parlamento, vorrei estendere il mio apprezzamento anche al ministro D'Incà. So che quello del MES era ed è un tema non facile per il MoVimento 5 Stelle; non facile, ma - lo penso da tempo - non impossibile. Sedendo in questa posizione qui in Senato, circondato da senatori del MoVimento 5 Stelle, mi sono fatto impressioni e percezioni - qualche volta si ascolta anche senza volerlo - che il MES non era un argomento impossibile.

Questo impegno mi sembra che finalmente sia avvenuto e abbia dato i suoi frutti, consentendo persino a una forza che si presentava con connotati così diversi al momento della sua apparizione in scena di scoprire che non aveva proprio niente contro l'Europa. *(Applausi).* Ebbene, credo che lei abbia fatto bene a non forzare chiedendo chiedendo oggi anche l'autorizzazione all'utilizzo del MES sanitario. Ripeto: credo che abbia fatto bene. Sono però tra coloro che pensano che lei dovrebbe fare presto questo secondo passo. Perché non avviene questo? Intuisco due possibili motivi di *Realpolitik* poco confessabili, e sento parlare invece di un motivo, quello dello stigma, secondo me non reale.

Io la chiamerei una benedizione, perché in Italia il sistema sanitario con le sue forze non ha la capacità di generare in questa e nell'altra Aula consenso per 37 miliardi. Ma se proprio devono essere destinati a questo, i 37 miliardi verranno destinati a questo. Altro motivo per cui forse si rilutta è che i soldi del MES, per i quali lo Stato si indebiterebbe, andrebbero alle Regioni, che in Italia gestiscono il sistema sanitario largamente e che non sono tutte necessariamente dello stesso colore politico del Governo. Io li chiamerei «motivi Ci si parla di stigma. Colleghi, permettetemi di essere franco: lo stigma, lo sfavore dei mercati, colpisce un Paese non perché fa uso di un certo strumento finanziario, ma per la politica ma per la politica economica e il Governo che quel Paese ha. Allora credo che convenga trarre qualche motivo di consolazione per il fatto che la misura dello stigma contro l'Italia, pur essendo ancora elevata, si è ridotta nel corso del tempo. tempo. Permettetemi però di dire che il vero stigma è che oggi, essendo a 120 punti lo *spread* dell'Italia, questo superi il 24 della Francia, il 31 dell'Irlanda, il 60 del Portogallo, il 64 della Spagna e il 76 di Cipro (Paese stigmatico per definizione, verrebbe da dire). Anche in tempi di tempeste finanziarie grandi, che molti di noi ricordano, lo *spread* dell'Italia è sempre stato sotto lo *spread* della Spagna, oggi è il doppio. Questi sono gli stigmi a cui dedicare attenzione, secondo me. Concludo dicendo che anch'io, come tutti, sono interessatissimo a quello che lei, signor Presidente, presenterà in materia di Piano nazionale di ripresa e di resilienza. Due note soltanto: credo si tratti di ravvivare la pubblica amministrazione attraverso l'assunzione di giovani qualificati, non di creare - come si fa con le imprese a volte - una *bad* PA e accanto una *good* PA. In secondo luogo, si tratta anche di stimolare la concorrenza e di combattere le rendite di posizione, cosa che credo farebbe molto piacere che sono entrate in questo Parlamento nel 2018. Questo non lo si farebbe estendendo l'ala di chi dirige imprese pubbliche al resto dell'economia, creando anche molti possibili conflitti.

chiedendo deroga al mio Capogruppo o a chi di dovere. Su tutte le partite dei fondi europei ho serie riserve. Rendo onore a chi votò no al *fiscal compact* nel 2012: al senatore Vitali, allora deputato, e al mio amico Guido Crosetto, perché erano previsioni inattuabili, non si potevano votare, tanto che oggi sono sospese. L'Italia risulta avere già versato 14,1 miliardi al MES e ha un impegno pluriennale fino a 125 miliardi, che corrispondono alla sua quota del 17,7. Sotteso a questi discorsi - come a tanti altri dell'Europa - c'è la cessione di sovranità all'Europa. In tema Macron, due giorni fa, ha abbracciato al-Sisi e del caso Regeni se n'è fatto un baffo, ammesso e non concesso che noi dobbiamo fare la guerra per Regeni. dell'economia: le banche tedesche e francesi sono piene di derivati, hanno dei problemi. L'acquisto delle nostre aziende è a prezzi di realizzo, ma provate ad acquistare un'azienda francese? Questa è la solidarietà europea. I diritti civili: l'eutanasia che ci predica l'Olanda, una società senza radici, senza storia, senza principi. Come avete finanziato gli scostamenti finora approvati fino a 108 miliardi? Con debito pubblico, con l'idea di applicare successivamente il meccanismo della sostituzione, cioè destinare i fondi europei senza aumentare troppo il debito. I fondi europei sono tutti debiti, sono scritti agli atti, basta leggerli per intero: anche gli 80 miliardi del *recovery fund* sono sussidi che, qualora non rimborsati o non rimborsabili, saranno sostituiti da tasse tasse europee (sull'ambiente, sulle transazioni finanziarie) oppure da un aumento del contributo annuo da parte di tutti i soci, se accetteranno, ma sarà il nostro contributo futuro ad aumentare. io ho letto così. le differenze di tasso sul MES, è il mercato che decide. Credo che si sia spiegato bene: il tasso sul BTP può diminuire. Può il MES, con i nostri soldi versati, prestarceli e poi chiedere delle condizioni? Sì, è scritto. Con la Grecia era un'altra fase, ma la vendita degli *asset* immobiliari - l'aeroporto, per citarne uno - e altri di tutta la poca industria della Grecia a prezzi di realizzo a cura della *troika* un caso di non restituzione. Si potrà applicare in Italia, eventualmente anche per fare altre spese fantasiose e infruttifere, tipiche di questo Governo, la patrimoniale. Ne avete parlato, poi avete fatto retromarcia, ma se ne avete parlato è perché comunque è nelle vostre intenzioni. Il MES, così com'è costituito, ha privilegi assurdi nella sua sostanza costitutiva; è oltre la legge.

solo inviolabili come persone e i loro domicili, le controversie le decidono loro: tutto a porte chiuse. Vi metto tutto sul piatto: come può il centrodestra sostenere e votare sì a queste condizioni in cui viviamo in questi tempi? Tralascio volutamente - perché non è argomento di oggi - la gestione della pandemia. L'ha accennato prima lei, Presidente, quando ha parlato della Libia: i pescatori sono ancora là, ma per i precedenti ostaggi si è pagato 10 milioni cadauno. Evito di fare i nomi per rispetto. *(Applausi)*. Ma visto che mi piace approfondire i temi economici, chiedo se i giacimenti di gas naturale e di petrolio dell'Adriatico

farne una sola pubblica; che bello, quando abbiamo impiegato vent'anni a farle diventare private. Per sicurezza, qualora ciò non avvenisse, avete già catapultato Padoan da deputato, eletto a Siena, direttamente a Unicredit per fare il presidente

nomina dei commissari per le opere pubbliche, le ricordo la nomina del commissario per il traforo del Colle di Tenda, in provincia di Cuneo, e la ringrazio anticipatamente. Che fare dunque? Prestito Prestito nazionale, redimibile o irredimibile: basta presentarlo bene agli italiani. Io parlo con la gente comune che mi dice: se dovessi versare mille euro e fossi sicuro che tutto va a buon fine lo farei; se dovessi sottoscrivere il debito pubblico...

Signor Presidente, colleghi senatori, presidente Conte, per me è un'emozione poter parlare oggi, perché penso a tutti i milioni di italiani che vorrebbero dirle qualcosa in questa giornata, soprattutto in questo periodo, dopo che è uscito l'ultimo decreto recepito con grande stupore. A Natale, nei giorni di festa, saremo tutti contingentati all'interno del nostro Comune, signor presidente Conte. Magari, se sta un attimo attento, senza guardare il telefonino; non so se ha

non so se a queste persone hanno pensato anche tutte le *task force*, che mi sembra siano una quindicina. Quindici *task force*, oltre mille consulenti, per partorire un DPCM del genere: mi sembra veramente gran poca cosa. Quindi, il mio augurio va a tutte quelle persone

Conte, distragga qualcuno di quegli agenti per scortare Brumotti quando va a indagare sugli spacci della droga, perché se ne va sempre da solo e le assicuro che in questo Paese di spacciatori di droga ne abbiamo tantissimi. Qualcuno lo mandi pure là.

per questo Paese. Qui occorre fare una riflessione: lei porterà l'esperienza ambientale dell'Italia, che si confronterà con quella dell'Inghilterra. Ma sappiamo che l'Inghilterra, dal punto di vista ambientale ha fatto

abbiamo investito 120 milioni di euro per comprare i giocattoli all'ex ministro Toninelli e a pochi altri fortunati italiani.

potrebbe dire al ministro Costa di dare questi 120 milioni di euro magari a tutti quegli agricoltori di montagna che non hanno più i soldi per andare avanti e stanno abbandonando il territorio. Sarebbe buona cosa poter conservare il territorio

spero che questo Natale non si permetta di fare gli auguri agli italiani, perché credo che gli italiani, dei suoi auguri di buon Natale, quest'anno se ne faranno ben poca cosa.

in questi giorni molti osservatori si sono esercitati nel presentare l'appuntamento odierno con le comunicazioni del Presidente del Consiglio, travisandone gli obiettivi. Innanzitutto dobbiamo concentrare la discussione sul vero tema del Consiglio europeo, ovvero arrivare in tempi rapidi allo sblocco delle risorse del *recovery fund*, fondamentali per il rilancio del Paese. In secondo luogo, si affronterà la modifica del MES, meccanismo già esistente dal 2012, approvato e avallato nel corso del 2011, dall'allora Governo di centrodestra, sostenuto dalla Lega e da diversi esponenti di quello che poi sarebbe diventato il partito Fratelli d'Italia. Questo per mettere in chiaro, una volta di più, chi ha fatto cosa a proposito del MES. Questa modifica del Trattato ha sicuramente luci e ombre. Tra gli aspetti positivi, ottenuti anche grazie all'impegno del Governo italiano, c'è l'anticipo al 2022 del cosiddetto *common backstop*, ovvero la possibilità che le risorse del MES sostengano il Fondo di risoluzione unico per le banche. Grazie al negoziato condotto dall'Italia si è potuta fondare la condivisione dei rischi associati al *common backstop* sul presupposto della netta riduzione dei rischi, operata da parte delle banche italiane, fino all'arrivo della pandemia. Ma la nostra posizione sul MES e quindi sul suo utilizzo non si è mossa di un millimetro. Noi del MoVimento 5 Stelle riteniamo questo istituto profondamente contrario ad una vera logica eurounitaria. Per noi il MES è anacronistico e improponibile in un'Unione europea, che nella nuova fase storica, apertasi dopo il Covid, ha già cominciato a cambiare sotto i nostri occhi, adottando finalmente soluzioni solidali e inclusive. Certo, queste soluzioni ancora non bastano; alcune sono ancora in corso di definizione, a cominciare dagli altri elementi del pacchetto di riforme dell'unione economica e monetaria che accompagnavano la riforma del MES, primo fra tutti uno schema di assicurazione europea sui depositi bancari (EDIS), che è l'elemento mancante per completare realmente l'unione bancaria. prima di un'eventuale ratifica della riforma del MES che dovrà essere effettuata dal Parlamento, ci riserveremo di valutare se vi siano stati davvero dei progressi adeguati e comprovati sugli altri elementi del pacchetto di riforme Continueremo ad essere vigili nella consapevolezza che non vi possano essere avanzamenti soltanto sulla parte del pacchetto senza che ve ne siano sull'intero percorso riformatore, ma proprio per questo riteniamo importante consentire al *premier* Conte di trattare in Europa un quadro complessivo di riforme indispensabili al futuro dell'Unione. oggi ha giustamente ha detto il presidente del Consiglio Conte nelle sue comunicazioni, la posta in gioco per costruire un'Europa profondamente diversa dal passato è ben più alta rispetto a tutte le questioni discusse prima dell'arrivo del Covid-19, compresa la riforma del MES. La crisi pandemica ha dimostrato in modo inequivocabile che l'unica possibilità per l'Unione europea e l'unione monetaria è quella di costruire istituzioni sempre più federali, dotate di una capacità di bilancio comune, che sappiano indicare le grandi priorità su cui tutti i Paesi europei dovranno investire con spirito di coesione e unità. Il modello del *recovery fund* costituisce l'esempio virtuoso da seguire in questo senso e va anzi reso strutturale, come ha ribadito il Presidente del Consiglio. Accanto ad esso va rafforzato il ruolo della Banca centrale europea a tutela della stabilità finanziaria e della crescita dell'eurozona, e vanno riviste radicalmente delle regole di bilancio la cui inadeguatezza è ormai sotto gli occhi di tutti. Vorrei ribadire ancora una volta che per quanto ci riguarda con il MoVimento 5 Stelle al Governo non c'è alcuna possibilità che l'Italia acceda ai prestiti del MES, una vera e propria spada di Damocle sulla testa del nostro sviluppo e delle future generazioni Tornando alla discussione all'ordine del giorno, essa appare troppo spesso viziata da sterili e strumentali tifoserie, lontane dalla necessità di concentrarsi su una seria proposta per portare il Paese fuori dalla crisi e proiettarlo nei prossimi decenni. Dispiace che a introdurre questi litigi sia stato, tra gli altri, anche qualche ex Presidente del Consiglio, più propenso disperdere energie nella gestione del proprio *ego* e dei suoi marginali calcoli politici, che nella risoluzione dei problemi del Paese. Poco male visto che a Palazzo Chigi oggi c'è chi, con il supporto del MoVimento 5 Stelle, sta cercando di innescare un cambiamento epocale nelle istituzioni europee, perché un'emergenza come quella del Covid-19 ha mostrato tutti i limiti delle politiche economiche adottate in precedenza Non basta una campanella a fare un Presidente del Consiglio. Giuseppe Conte ha da subito dimostrato, con le sue capacità, di essere all'altezza del nuovo corso e lo ha sempre fatto, fin dall'inizio della crisi pandemica, con grande responsabilità e soprattutto con estrema trasparenza. Vorrei ricordare a tutti il motivo per cui siamo qui in quest'Aula, cioè risolvere i problemi e disegnare un futuro per il Paese. Non può e non deve essere ridotto tutto a un sì o no al MES e alla sua riforma; si tratta di disegnare un quadro molto più vasto per i nostri figli. Il piano europeo per la ripartenza, infatti, si chiama Next generation EU e questo nome è stato scelto proprio perché il piano deve essere diretto alle future generazioni e non deve essere solo limitato al superamento delle contingenti difficoltà economiche e della crisi. In conclusione, è a questo quadro d'insieme che dobbiamo guardare; un quadro fatto finalmente di titoli di debito comune per finanziare il *recovery fund,* con la prospettiva di renderlo stabile, di stimoli monetari finalmente espansivi da parte della BCE, dell'apertura di un dibattito sulla modifica del Patto di stabilità dopo la sua ovvia sospensione. Lasciatemi dire che non occorrono personaggi legati alla prima Repubblica che somigliano - utilizzando una metafora cinematografica - a quel cacciatore di taglie che disse qualcosa del tipo: ehi tu, lo sai che la tua faccia somiglia a quella di uno che vale 2.000 dollari? Sì - gli riposero - ma tu non somigli a quello che li incassa. A voi tradurre la metafora. Rispetto al punto di partenza (marzo 2020) molta strada è stata fatta e noi siamo qui per permettere al Presidente del Consiglio di farne tanta altra. Presidente del Consiglio Conte, lei è una brava persona e in quest'Aula ho sofferto a vedere come la critica politica, ovviamente permessa per carità, si sia trasformata spesso in dileggio verso la sua persona e l'operato del Governo. Oggi che ho la possibilità di contrastare questo comportamento per me inaccettabile, lo faccio senza indugio e le rinnovo stima e fiducia anche livello personale.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

È sicuramente propaganda da campagna elettorale, è tutto strumentale. Il MES esiste da dieci anni e per poter esserci l'Italia ha versato anche diversi miliardi. La riforma non implica nuove spese e non pone nuove condizionalità; non comprendo perché si sia insinuato nei giorni scorsi tra alcune forze politiche il giudizio apodittico sulla presunta inadeguatezza di questa linea di credito per il nostro Paese, che spesso è stato ripetuto senza essere accompagnato da una qualche analisi rigorosa. Non la pensa così infatti la Banca d'Italia e non la pensano così i maggiori economisti; meno male che alla fine sia prevalso il buon senso. Le ragioni del no al MES avrebbero creato sconcerto nelle cancellerie europee data la palese dimostrazione dell'incapacità di saper vivere momenti storici privi di cipiglio ideologico e di strumentale resa dei conti. Il punto di caduta finalmente si è avuto; abbiamo evitato la brutta figura, ma così facendo si apre sempre più una voragine tra noi e il Paese. Forse la gente inizia, signor Presidente, a pensare che prima del vaccino anti-Covid, occorra che la classe politica si faccia iniettare il vaccino del buon senso. Non si avvantaggiano le banche tedesche, come qualcuno ad arte sostiene, né faremo la fine della Grecia. Con il voto di oggi decidiamo il futuro insieme ad altri, stando ai patti che i vari Governi degli ultimi anni hanno sottoscritto. Governi ad immagine delle zone

Avrei auspicato così. In questa maggioranza nessuno pensi che noi siamo i sostituti delle beghe altrui, e non possono essere i colleghi del MoVimento 5 Stelle partito di lotta e di Governo; decidete il vostro destino perché noi non vogliamo dipendere dal vostro. La mia storia politica ha visto lotte di correnti, ma ideologismi e fumerie senza senso mai; no, mai. Per oggi la crisi pare scongiurata. Così però si fa fatica ad andare avanti e, soprattutto, crescono in giro collera e disappunto e il carro con le ruote quadrate, come ha detto il Censis, avanza a fatica, fatica, a stento. Certo, perché il carro vada veloce occorre che tutti si dia una mano, non solo oggi con il MES, signor Presidente, ma anche con il *recovery fund*. Il Parlamento recuperi perciò la sua centralità, mortificata da questa filiera istituzionale sfilacciata.

sono tra coloro che ritengono che lei, signor Presidente del Consiglio, abbia fatto la cosa giusta a procedere sulla strada tracciata dal ministro Gualtieri quando, settimane fa, ha dato il proprio consenso, il consenso del Governo che lei rappresenta, alla riforma del MES. Del resto si tratta di una riforma non assolutamente peggiorativa; del resto permanere in una posizione diversa avrebbe significato isolare il Paese che lei rappresenta e intralciare, profondamente intralciare, il cammino del *recovery fund*. Di nessuna utilità quindi. È la ragione per la quale è incomprensibile, tanto più se letto all'interno della grande casa del Partito popolare europeo, l'atteggiamento di Forza Italia, che ha tenuto e continua a tenere - ne sono assolutamente lieto e lo riconosco - una posizione di cornice assolutamente importante, ma incomprensibile proprio nel caso di cui stiamo discutendo. Al contempo, presidente Conte, la sua comunicazione non mi ha assolutamente rassicurato. di quanto sarebbe potuto accadere oggi: di un arsenale pronto a esplodere, ma che sicuramente - e lo sapevamo - non esploderà. Questo, Questo, però, non significa che il cammino non sia accidentato. Signor Presidente del Consiglio, mi sarei augurato che lei oggi in Aula, di fronte al Senato della Repubblica, più che parlare dei contenuti di merito del Consiglio europeo, avesse preso per le corna la testa del toro.

È accidentato perché oggi abbiamo la riforma del MES; domani abbiamo una gigantesca *task force*, sulla quale la mia opinione è nota (ma fra un po' la ripeterò); poi avremo il tema centrale del *recovery fund*; dopodomani avremo la questione di due Regioni non secondarie, come il Lazio e l'Emilia-Romagna, che chiedono di essere direttamente interessate dalla questione del *recovery fund*. In ultimo, ma non ultimo, rimarrà aperta la questione se questa straordinaria Italia utilizzerà o meno i fondi del MES. Non mi preoccuperei granché del rimpasto. C'è una sorta di rimpasto sotterraneo che prosegue da tempo, fatto di commissari che hanno appunto poteri straordinari. Se dovesse realizzarsi una *task force* di dimensioni elefantiache e mastodontiche, i Ministri verrebbero in qualche modo deprivati di funzioni primarie. Soprattutto, siamo di fronte a una sotterranea,

parliamo di una relazione apicale quasi esclusiva tra il Governo e i suoi vertici e le Regioni italiane, con Governatori che hanno ormai poteri superiori a chi siede nell'Esecutivo. Concludo rapidamente, signor Presidente.

era lui che aveva bisogno di dimostrare fiducia agli italiani. Questa non è la primavera: allora c'era speranza, oggi il rischio è apatia e rassegnazione. Segua quella strada, coinvolga di più il Parlamento, usi di più l'articolo 120 della Costituzione quando c'è da dipanare una matassa difficile con le Regioni e deliberi rapidamente l'accesso al MES. Risparmiamo poco? Sono 300 milioni. Abbiamo salutato 50 milioni di risparmio per il taglio dei parlamentari come se ci fossimo arrampicati sulla luna. Qui sono 300 milioni. Andiamo sul libero mercato a cercarli? Lo faremo fra poco, perché

salvo qualche colpevole omissione per quanto riguarda, ad esempio, il terrorismo islamico, che è spesso anche importato più di quanto non sarebbe necessario. Noi, invece, abbiamo scelto di presentare una risoluzione sul problema che ci sembrava più ostico e difficile da risolvere, che è all'ordine del giorno dell'Eurogruppo e non anche del Consiglio dei Capi di Governo e di Stato. È un problema difficile perché, a mio avviso, c'è anche una considerazione iniziale che possiamo fare. Tutti gli strumenti europei tendenzialmente, ma soprattutto il MES nel nuovo ruolo che viene ad assumere hanno fondamentalmente una funzione di deterrenza nei confronti di eventuali speculazioni che possono avvenire sui mercati. Tutti ricorderanno la famosa frase che fu pronunciata dal presidente Draghi nel 2012 quando disse: «*Whatever it takes*». Lo poté dire - fu possibile per lui enunciare quella frase - perché la richiesta di aiuto

L'effetto deterrenza funzionò a meraviglia perché non fu poi obbligatorio utilizzare quello strumento. Alcune modifiche vanno sicuramente nella direzione della maggiore deterrenza dello strumento europeo che viene adottato; altre sono, invece, modifiche sostanziali

il problema è che bisogna fare un *memorandum of understanding* (MOU) in una trattativa fra lo Stato, la Commissione europea, il MES e in questo caso anche il direttore generale del MES. importante modifica è, infatti, proprio il ruolo del direttore generale, che diventa importante nella misura in cui si sposta l'asse del potere politico dalla Commissione europea per questi problemi al MES. il MES sarebbe dovuto diventare un fondo monetario europeo, ma non fu possibile arrivare a questo accordo ed è rimasto un'associazione intergovernativa.

Ci sono tre modalità di voto del MES: c'è il voto all'unanimità, c'è il voto al 85 per cento, che viene attivato nel momento in cui c'è un provvedimento di urgenza da prendere e c'è il voto all'80 per cento per il direttore generale del MES.

Il terzo pilastro della riforma è il *backstop*, una specie di paracadute che viene fornito dal MES al Fondo di risoluzione unico. Come ben sapete, il Fondo di risoluzione unico ammonta a circa 60 miliardi, una provvista fornita dalle banche e dalle istituzioni finanziarie. Questo paracadute - questo sì, come dicevo prima - ha un effetto di deterrenza importante perché, ove dovesse verificarsi un possibile *default* di una banca e di un sistema bancario, per evitare il contagio potrebbe intervenire prima il Fondo di risoluzione unico e poi la garanzia del paracadute fornito dal MES.

la possibilità di bloccare i patti di stabilità - oltre alla considerazione sugli aiuti di Stato, che venivano resi possibili - e c'è stato fondamentalmente il grande cambiamento del paradigma di fondo del sistema economico europeo, con la mutualizzazione del debito, che produrrà le risorse per il *recovery fund*, mi rendo conto della difficoltà che lei potrà avere in Europa ad assumere una posizione di forte critica rispetto ad un accordo che, per certi versi, era già stato preso nel 2019. Le motivazioni che ci hanno dato lo spunto per presentare una risoluzione sono dunque abbastanza semplici e voglio richiamarle con chiarezza. La prima, si sostanzia nel fatto che nella definizione della divisione di ruoli tra la Commissione europea e il MES riteniamo sia necessario un maggiore chiarimento, in particolar modo escludendo l'affidamento al MES di compiti di sorveglianza macroeconomica sarebbe anche una duplicazione rispetto alle competenze della Commissione europea. La seconda motivazione riguarda la valutazione di quei prerequisiti di cui parlavo prima per la possibilità di accesso alle PCCL, che invece dovrebbe trasformarsi in una considerazione generale della situazione macroeconomica del Paese richiedente. Il terzo motivo, molto importante e del quale non ho ancora parlato, è che si debba e si possa escludere in ogni caso ogni meccanismo automatico di ristrutturazione dei debiti sovrani.

ovviamente come Gruppo Misto Idea e Cambiamo non possiamo assolutamente votare la risoluzione della maggioranza che, per quanto riguarda il MES, propone un compromesso al ribasso, chiaramente frutto dei conflitti e delle difficoltà

Conte, perché la discussione che ha preparato questo incontro e le sue comunicazioni, questa mattina alla Camera e oggi pomeriggio qui in Senato, è stata scandita da un'attenzione solamente ad uno dei

Proprio in questi giorni siamo dinanzi a inondazioni, alluvioni, frane, smottamenti, tempeste, acqua alta a Venezia. Se non interveniamo, è del tutto evidente che sarà ancora peggio di così. Avremo - e abbiamo già - impatti devastanti sull'ecosistema, sulle migrazioni, sull'economia, sulla lotta per le risorse e sulla pace nel mondo. il tema che lei domani andrà a dibattere a nome di tutti gli italiani, relativo al cambiamento climatico - il secondo punto all'ordine del giorno - parla esattamente di questo, di una questione di straordinaria importanza per il nostro presente e per il nostro futuro. Va riconosciuto che l'Unione europea in questa direzione non è stata ferma. Il primo pacchetto - come è noto a chi legge almeno qualche carta - è del 2008 e ha fissato gli obiettivi che, guarda caso, scadono proprio nel 2020, cioè, relativamente

Nel dicembre 2019 i *leader* europei hanno approvato l'obiettivo di raggiungere l'impatto climatico zero nel 2050, ma la Polonia si è opposta; guarda caso ancora la Polonia, anche su questo tema. Da lì è nato tutto un grandissimo lavorio. A caduta, nell'ottobre 2020, il Consiglio europeo ha discusso la comunicazione della Commissione sul tema del nuovo traguardo della neutralità climatica

anche gli europarlamentari della Lega, di Fratelli d'Italia e la gran parte dei parlamentari di Forza Italia. Esattamente l'opposto della nostra risoluzione, che invece va nella direzione di accogliere e di spingere

Dicevo prima che l'Unione europea non è stata ferma. Abbiamo introdotto nel nostro ordinamento, attraverso leggi che abbiamo votato anche in questo Senato, il pacchetto dell'economia circolare nel maggio 2019, il pacchetto energia pulita, la diminuzione delle emissioni di CO2 nei trasporti, in particolare con la regolamentazione della gomma nell'aprile 2019. C'è poi tutto il sistema di scambio delle emissioni nell'Unione europea, che sta creando il più grande mercato mondiale del carbonio nel nostro continente. Bene, signor Presidente, se questo è esattamente quello che è stato fatto in questi anni, ora è del tutto evidente che la grande sfida nel medio periodo è quella della pandemia. Non c'è dubbio alcuno sul fatto che la pandemia la si sconfigge con una visione panecologica, comprendendo che siamo un unico ecosistema. Ogni sovranismo è strutturalmente del tutto incapace anche solo di sillabare le soluzioni. D'altro canto, colleghi, quale sovranità nazionale chiusa e autoreferente può sconfiggere i temi all'ordine del giorno nel Consiglio di domani? Mi riferisco ai temi della pandemia, del cambiamento climatico, della sicurezza e della lotta al terrorismo.

da alcuni anche in questo Parlamento voluti, o proseguiva con direzione convinta verso un processo di integrazione. Ha scelto la seconda strada. Presidente, a nome del nostro Gruppo, per quanto riguarda in particolare il tema *green*, andiamo avanti con questa grande determinazione, perché lo sviluppo non ci potrà essere se non sarà sostenibile dal punto di vista sociale, economico e ambientale.

Lo facciamo in maniera molto convinta, dopo esserci prodigati in queste settimane a cercare di spiegare alle tante persone che ci vengono incontro che cosa significa questo grande dibattito sul MES, che a un certo punto sembrava volesse spaccare la maggioranza e anche addirittura porsi come un elemento di criticità rispetto alla tenuta del Governo. Quando ci siamo espressi con una chiarezza assoluta sul fatto che noi avremmo votato a favore della riforma del MES - e lo spiegherò, spero, con sufficiente chiarezza qualcuno ha pensato che volessimo fare da stampella al Governo. Abbiamo in proposito ribadito più di una volta che non avevamo nessuna intenzione di fare da stampella al Governo, anche perché, molto probabilmente, il Governo non avrebbe avuto bisogno di una stampella dal momento che, davanti al rischio di precipitare, molte persone si sarebbero ravvedute e, all'interno della stessa maggioranza, avrebbero votato a favore. per noi era importante votare a favore della riforma di questo Trattato, perché quello precedente di fatto ha segnato in modo drammatico il destino della Grecia,

quasi persecutorio; la stessa Merkel è tornata molte volte a denunciare gli errori che l'Europa stessa aveva commesso nei confronti della Grecia con quel trattato,

subordinata a un grande progetto sociale, inclusivo e capace di valorizzare le nuove generazioni (non a caso il *recovery fund* in altri posti si chiama New generation EU ed è orientato a togliere dalle spalle delle nuove generazioni una sorta di capestro e a liberarne la creatività, lo spirito di iniziativa, la voglia di riappropriarsi del loro futuro)

ci piace. Noi vogliamo la riforma del Trattato perché vorremmo davvero, con grande intensità, che il Governo attingesse alle risorse del MES;

potremmo disporre di 37 miliardi di euro orientati alla salute dei cittadini, dall'altra parte sappiamo bene che ce ne sono scarsamente nove di miliardi, del tutto insufficienti ad avviare il processo di riforma che auspichiamo.

e dai nostri alleati della Lega, che sono contro la riforma e contro le risorse. Ma noi siamo noi; siamo una grande e antica struttura di centro, con la propria visione della società, con la propria visione economica, con la propria visione culturale ed è quella che vogliamo riaffermare oggi, con il nostro voto favorevole al MES, ma contrario alla risoluzione del Governo, che, come è stato detto dal mio collega pochi minuti fa, affoga in dieci pagine in dieci pagine una riga e mezza in cui parla del MES: evidentemente hanno faticato molto a trovare il loro punto di convergenza. Su questa fragilità del punto di convergenza evidentemente si costruiranno ulteriori soluzioni a rischio, con cui il Governo continua a oscillare, tra Scilla e Cariddi, tra gli uni e gli altri. Noi crediamo che gli italiani meritino qualcosa di più; crediamo davvero che agli italiani debba essere dato uno strumento di garanzia chiaro, forte e potente, che non sia una dialettica meramente ideologica, ma una presa di posizione importante al servizio esclusivo della loro salute, per tutte quelle iniziative che abbiamo tante volte ricordato anche al ministro Speranza. Noi vorremmo davvero che questa fosse la volta buona, in cui gli specializzandi della facoltà di medicina, gli anziani disabili e le persone con criticità possano trovare quella famosa assistenza socio-sanitaria verso cui abbiamo bisogno di spostare l'asse: dalla struttura ospedaliera alla struttura del territorio. Noi vogliamo una ricerca molto più forte. Nella legge di bilancio c'è pochissimo per la ricerca. la ricerca. E la ricerca non è solo la ricerca del vaccino. Esiste anche la ricerca sui farmaci rari, la ricerca è anche orientata a promuovere nuove forme di salute e nuove risposte ai bisogni emergenti. In tutto questo, ci piacerebbe poter ribadire che il nostro no si estende anche alla cabina di regia extraparlamentare che in qualche modo offende e umilia l'intero Parlamento.

la prima domanda che mi sono posto all'inizio di questo dibattito è: a chi giova? *Cui prodest*? È evidente, infatti, che se c'è una votazione, se c'è un voto, ci deve essere anche un interesse legittimo che deve essere perseguito. La prima risposta potrebbe essere che giova al Paese, ma non credo. Il dibattito e anche il dissanguamento che abbiamo visto nei giorni scorsi sulle pagine dei giornali da parte del MoVimento 5 Stelle, come anche come anche lo *scouting* che sta avvenendo, ancora in queste ore, qui fuori, oltre alle assenze per malattia che avremo al momento della votazione ci dicono che la questione ha ben altre radici.

sera» che contiene la risposta. A chi giova? A chi serve questa votazione? Serve al Paese? No, questa votazione serve esclusivamente al manovratore per poter continuare ad andare avanti. a colui che, oggi molto distratto, un tempo si presentò in quest'Aula dicendo di essere l'avvocato degli italiani, l'avvocato del popolo. Ma è evidente che, come dice il presidente Fico, tutto deve essere fatto in funzione del permanere di Conte alla Presidenza del Consiglio dei ministri, poco importa il merito e poco importa il contenuto. Importa talmente tanto poco

Presidente, è che oggi pochi hanno la possibilità di essere veramente liberi e di poter dire no, perché dire no significa anche ridare la voce ai cittadini, ad esempio, significa magari prendere una posizione che ti porti in contrasto con il tuo Gruppo, se sei veramente libero dal vincolo di mandato e fai quello che serve al popolo, non quello che serve a Casaleggio. Il problema, però, si pone perché nel momento in cui la retorica 5 Stelle ha continuato a minare alle basi le fondamenta della nostra democrazia, oggi in questa sede - e mi spiace, purtroppo, perché c'è anche gente seria che rispetto ci troviamo con tanti parlamentari che se dovessero tornare a casa sarebbero costretti a compilare immediatamente il foglio per il reddito di cittadinanza. Quando si è trattato di staccare la spina della maggioranza, noi l'abbiamo fatto senza pensare al nostro interesse, ma pensando innanzitutto al bene del Paese. Oggi, invece, ci viene detto che tutto va bene, ciò che importa è che Conte stia in piedi. Ma allora mi domando perché nel vostro eccesso di democrazia questa volta «Rousseau» lo avete lasciato nel cassetto? Perché non siete andati a chiedere ai vostri iscritti cosa ne pensano del MES? Perché questo lo fate solo quando vi conviene, solo quando siete sicuri che l'esito che esce da quella votazione sia quello che fa comodo al manovratore. Ben ve ne guardate, in questo momento, di ricorrere a quella stessa democrazia partecipata con cui vi siete sciacquati la bocca. Noi possiamo dire oggi che eravamo contrari

voi non potrete più farlo perché oggi tradite voi stessi e il vostro elettorato. La distanza che si è creata nel Paese non è solo la distanza tra voi, la gente che vi ha votato e il resto del Paese, ma è anche una distanza che si è creata tra chi sta ai piani bassi e chi sta ai piani alti. Voi qui, infatti, oggi fate solo quanto serve al manovratore che sta al Governo Governo e quanto serve per mantenere certi Ministri al Governo, magari quelli che hanno dovuto cambiare due Ministeri e che sono pronti, come è già stato in altre epoche, a cambiarne anche tre, se serve, pur di restare al Governo. Questo è oggi il motivo che porta al vostro voto. So che non siete tutti piegati a questa

dell'Unione europea dice in maniera chiara e incontrovertibile che ci devono essere rigorose condizionalità. Badate bene, mettere sullo stesso piano una norma con una letterina che arriva da un commissario europeo non è la stessa cosa. Voi oggi, se fate la scelta sbagliata, metterete un cappio al collo all'Italia, e hai voglia a dire che riformate quel cappio. *(Applausi).* Cappio è e cappio resta! Ancora una volta, a chi serve tutto questo? Serve al presidente del Consiglio Conte, perché, come dice il la maggioranza ha il dovere di sostenere Conte. Badate bene: non dice che ha il dovere di sostenere l'Italia e il Paese, ma di sostenere Conte, che è ben altra cosa rispetto al bene del Paese. *(Applausi).* Qui si confonde il singolo con l'interesse generale. E chi è questo signor Conte, l'avvocato Conte? È quello che il 30 gennaio diceva: «Eravamo già molto vigili e molto attenti nel monitorare l'evoluzione di questa situazione critica, non ci siamo fatti trovare impreparati»; «È tutto sotto controllo». E ancora il 26 marzo: «Nessuno resterà indietro». Lo abbiamo ben visto! Il 6 aprile: liquidità immediata per tutte le imprese; abbiamo messo in campo «una potenza di fuoco mai vista». Eccome, se l'abbiamo vista! ancora: «Abbiamo aumentato i posti in terapia intensiva»; «Tutto sotto controllo». Il 25 ottobre: «Chiudiamo tutto per salvare il Natale». Il 3 dicembre è andato in televisione a dire: tutti chiusi a casa a Natale. Questa persona non è credibile e non è credibile il suo Governo in Europa.

quanto fa Conte non va bene, e se Conte dice che va bene, dice solo delle gran balle. E il dovere importante che noi oggi abbiamo non è quello di tenere in piedi Conte, ma di tenere in piedi l'Italia!

grazie per le comunicazioni che ha reso, molto chiare, esaustive e condivisibili. Oggi è un giorno importante per il MoVimento 5 Stelle, perché segna una tappa significativa in quel percorso di cambiamento delle politiche europee che ci eravamo prefissi quando siamo entrati in Parlamento nel 2013. Volevamo superare le politiche di *austerity*, volevamo un'Europa solidale con i Paesi in difficoltà e non un'Europa matrigna; volevamo un'Europa non punitiva, che non imponesse sacrifici agli Stati momentaneamente in crisi e che non obbligasse a tagliare le pensioni, i salari i servizi essenziali quali la scuola, la sanità e la sicurezza. Volevamo una più profonda integrazione bancaria, che garantisse i depositi dei risparmiatori e non li esponesse ai disastri che hanno dovuto patire i nostri connazionali coinvolti nei *crack* di alcune banche italiane.

e priva di logica che ingessava e ingabbiava la nostra economia, impedendo a essa di crescere e di liberare tutte le sue enormi potenzialità. Infine, non volevamo un Meccanismo europeo di stabilità, che è nato come una sorta di banca, estraneo alle istituzioni dell'Unione, il cui *board* attualmente è formato da soggetti che nulla hanno a che fare con l'Europa. In buona sostanza, il nostro obiettivo era cambiare tutte le decisioni che in Europa e in Italia sono state prese, approvate e ratificate dal 2010 al 2012, sotto il Governo Berlusconi IV, sostenuto dalla Lega e dal Popolo delle Libertà, cioè da Forza Italia e da Alleanza Nazionale - cosa che oggi tutto il centrodestra

Cosa abbiamo ottenuto in questi mesi e nelle ultime settimane, in concomitanza della pandemia che ha sconvolto il mondo? Sostanzialmente cinque obiettivi: anzitutto, un piano pandemico di acquisto dei titoli di Stato da parte della BCE, prima stabilito in 750 miliardi, poi salito a 1.350 miliardi, e ora si parla di un'ulteriore espansione tra 500 e 600 miliardi; quindi, stiamo parlando di numeri assolutamente colossali, che hanno consentito al nostro Paese di mantenere basso lo *spread*; poi, il superamento di fatto di alcune regole di ingaggio, sempre della BCE, nell'acquisto dei titoli, come la famosa *capital key,* ovvero acquisti limitati in proporzione alla quota detenuta da una singola banca centrale nel capitale della BCE. Altro risultato importantissimo: la sospensione del Patto di stabilità, che di certo non potrà mai più essere come prima, perché siamo noi al Governo: questa è la differenza. Poi, la sospensione delle rigide regole agli aiuti di Stato, ma soprattutto abbiamo ottenuto un risultato fondamentale, che può davvero diventare un risultato storico nell'evoluzione europea. L'abbiamo raggiunto tra marzo e luglio di quest'anno, quando siamo stati capaci di convincere dapprima otto Paesi europei, e poi tutta l'Unione, a istituire il *recovery fund* (o Next generation EU, che dir si voglia), cioè, uno strumento completamente nuovo, dotato di 750 miliardi, per affrontare la crisi pandemica da Covid. Tale strumento si fonda, per la prima volta, su un debito in comune: un *recovery* che prevede per l'Italia, come è noto, fondi pari a 209 miliardi, 81 dei quali a fondo perduto. Altro che l'*austerity* del 2011, altro che la letterina della BCE che il 5 agosto 2011 *(Applausi)* arrivò al Governo Berlusconi, con la lista delle cose da fare per evitare il *default* dell'Italia, visti i risultati che quei signori che governavano il nostro Paese avevano ottenuto al Governo in quegli anni.

Il nostro obiettivo, come detto, era ed è portare avanti il processo riformatore dell'Europa, al fine di cambiarla per sempre e in meglio, modificandone l'architettura istituzionale ed economica. Con le altre forze politiche che sostengono il Governo ci siamo confrontati costruttivamente e con coraggio - gliene do atto e ringrazio per la disponibilità la lungimiranza dimostrata siamo arrivati insieme a decidere, e oggi lo mettiamo nero su bianco, che vogliamo cambiare profondamente anche il Patto di stabilità. Quindi, quella che prima era una logica di pacchetto che prevedeva tre elementi (la riforma del MES, accompagnata dall'EDIS e dal BICC, ovvero il bilancio della zona euro), ora ne prevede altri due, e cioè la profonda riforma del Patto di stabilità e le modifiche dell'architettura istituzionale economica dell'Europa, a cui facevo cenno prima, che si renderanno necessarie per costruire finalmente una nuova Europa, una nuova stagione dell'integrazione europea, che probabilmente va nel senso sognato dai Padri fondatori. Voglio sottolineare - e oggi lo scriviamo in modo chiaro e netto nella risoluzione che ci accingiamo ad approvare - che pretendiamo che lo stato di avanzamento dei lavori in merito alla riforma o alla costruzione di questi cinque elementi che compongono il pacchetto dovranno procedere di pari passo e il Parlamento dovrà verificare che tutto vada in tal senso, prima della ratifica parlamentare della modifica del Trattato del MES: questo per noi è irrinunciabile. A proposito del MES, devo dire che in questi ultimi mesi e anche oggi in Aula abbiamo assistito a una campagna di disinformazione indegna da parte dell'opposizione. Da marzo in poi non è passato un solo giorno senza che Salvini, Meloni ed altri raccontassero la menzogna che Conte aveva firmato o richiesto il MES nottetempo. A volte dicevano «firmato», a volte dicevano «richiesto»; non avevano nemmeno le idee ben chiare. Invece, la verità storica, scritta nei Resoconti delle Camere e della Presidenza del Consiglio, nelle carte ufficiali, nei libri di storia e in quelli di cronaca, è che il MES è stato approvato dal Governo Berlusconi IV, con dentro la Lega e il centrodestra,

alle ore 10,50 (vi posso dire anche l'ora a cui vi siete riuniti), il Consiglio dei ministri di quello stesso Governo Berlusconi... *(Commenti)*. Lo so che vi dà fastidio che vi ricordi queste cose, le vostre magagne. *(Applausi. Commenti)*. Purtroppo mi dovrete ascoltare; siamo ancora in democrazia, quindi mi farete la cortesia di ascoltarmi.

Il Consiglio dei ministri del Governo Berlusconi IV, sostenuto convintamente e con forza dalla Lega, un Governo che aveva come Ministri, per esempio,

Era, lo ricordo ancora una volta, il 3 agosto 2011: l'avete approvato voi. *(Applausi)*. Quel Governo approvò quel disegno di legge, perché, tra l'altro, il MES era uno strumento che combaciava perfettamente con le loro convinzioni politiche ed economiche, che i vari Tremonti e Brunetta ci raccontavano ogni sera in TV. Mi avvio a concludere: noi oggi non noi oggi non approviamo il MES per la semplice ragione - come ho cercato di spiegare - che lo approvò il centrodestra prima con la Lega dentro e poi con Monti tra il 2010 e il 2012.

non ne richiediamo il finanziamento, perché finché ci sarà il MoVimento 5 Stelle al Governo la linea di credito del MES non sarà mai richiesta dall'Italia, perché non ne abbiamo bisogno. Infatti, non abbiamo necessità di cassa, come affermato dal ministro Gualtieri qualche settimana fa, perché riusciamo a finanziarci benissimo sui mercati, tant'è vero che ormai paghiamo tassi negativi o pari allo zero per titoli fino a sette anni. Concludo: oggi, approvando questa risoluzione, ribadiamo la centralità del Parlamento nelle scelte strategiche di politica economica e facciamo un passaggio fondamentale nel percorso di riforma economica e politica dell'Europa, percorso che al suo termine vedrà un'Unione più equa, più giusta, più solidale, più lungimirante, più solidaristica e più vicina ai cittadini europei. Noi del MoVimento 5 Stelle ne siamo profondamente orgogliosi e allo stesso tempo siamo grati a tutte le forze politiche... Ha già concluso, per cortesia. Lei ha sforato di più di due minuti. Avevo raccomandato di attenersi ai tempi e lei ha sforato per più di due minuti. Siamo grati a tutte le forze politiche che in Italia e in Europa sono al nostro fianco in questo ambizioso progetto. Buon lavoro, Presidente.

signor Presidente del Consiglio, qualsiasi osservatore esterno direbbe oggi che il dibattito sul MES in Italia è più che strano: ha dell'assurdo. Il punto vero è che questo dibattito nasconde una vecchia questione, che non è un tema di maggioranza o di opposizione, ma è la linea di frattura tra chi crede nell'Europa e chi nell'Europa non vuole credere. Come autonomisti e come rappresentanti di una terra che, grazie all'Unione, è riuscita a sanare le ferite della propria storia, apparteniamo convintamente ai primi e vi apparteniamo da sempre, non solo da quest'anno, in cui l'Europa sta scrivendo una delle sue pagine più belle e importanti. Avevamo sperato che il *recovery fund* avesse definitivamente consegnato l'euroscetticismo alla storia, abbiamo peccato di ottimismo. In fondo, se c'è gente che, nel pieno di una pandemia, nega l'esistenza del virus, perché non credere ancora nel ritornello dell'Europa cattiva e pronta a dettare le sue leggi all'Italia? Ci servirebbe un vaccino anche per questo, perché si tratta di un virus che fa parecchi danni. Con questo non voglio dire che l'Europa sia la migliore delle istituzioni possibili. C'è ancora tanto da fare, sul fronte dell'integrazione fiscale e di una politica estera e di difesa davvero comuni, con una riforma della *governance* che aumenti il peso specifico del Parlamento europeo e porti ad un nesso più stringente con l'operato della Commissione. per superare veti e diffidenze, guidati dall'idea che cedere una parte della sovranità permette di guadagnare forza e influenza nelle sfide economiche e politiche dello scenario globale e questo anche attraverso il consolidamento della sussidiarietà in grado di valorizzare gli enti di prossimità, come le Regioni e i Comuni, che meglio possono rispondere alle esigenze immediate dei cittadini. Dovremmo discutere di questo, di come rilanciare questi obiettivi, nel contesto di una nuova primavera europea, cui la riforma del MES è soltanto un tassello e forse neanche quello più importante. Mi colpisce la difficoltà con cui la maggioranza è riuscita a trovare una mediazione e mi colpisce anche la posizione assunta da quelle forze d'opposizione, che fino all'altro ieri si professavano europeiste. Allora oggi guardiamo il bicchiere mezzo pieno, perché l'Italia rischiava di dare un duro colpo all'avvio di questa nuova stagione, che ancora si scontra con l'opposizione di Polonia e Ungheria. Guardiamola così, senza dimenticare che la riforma del MES porta delle migliorie, che vanno incontro alle esigenze italiane. L'Italia, infatti, non può annoverarsi tra i Paesi a rischio *default* e guai se qualcuno in quest'Aula lo pensasse. È vero che il nostro debito è pesante, ma l'Italia è una delle più importanti economie dell'eurozona e ha dalla sua un tessuto produttivo ricco e articolato. È il Paese con le maggiori potenzialità di crescita, se saprà riformarsi - penso alla pubblica amministrazione, alla giustizia e all'evasione fiscale

potrebbe essere nel sistema bancario, per via della durissima crisi che tutti stiamo attraversando e il fatto che ci sia un'assicurazione comune è positivo. Qualcuno dirà che così potremmo pagare il fallimento di una banca tedesca o francese, ma dico che non è importante se un euro italiano dovesse andare a queste banche, ballo c'è la tenuta di un disegno comune, in cui i benefici saranno sempre maggiori dei costi, come abbiamo visto in tutti questi mesi, grazie alla BCE. Inoltre, l'entrata in vigore del *backstop*, con due anni di anticipo, non vuol dire soltanto due anni di garanzia in più, vuol dire che non sappiamo come si evolverà la situazione e quindi non è scritto da nessuna parte che le condizioni di oggi potrebbero essere le stesse di domani. C'è poi la norma contro gli attacchi speculativi rivolti contro i Paesi sull'orlo del *default*. Non riguarderà sicuramente l'Italia, ma coloro che agitano da sempre lo spettro dei grandi poteri finanziari non si rendono conto del regalo che fanno loro non accettando la riforma. Allora il bicchiere è mezzo pieno, perché si è rischiato di infliggere un duro colpo al processo di integrazione, che ha preso nuova linfa proprio in questi mesi. Quale messaggio avremmo mandato al mondo? Quanta benzina avremmo messo nel motore di tutti quelli che torneranno a dire che il sogno di un'Europa veramente unita è solo un'utopia? Non potevamo permettercelo, come non possiamo permetterci, nel pieno di una sessione di bilancio, di una pandemia, della più grave crisi economica dalla fine della Seconda guerra mondiale, che si apra la stagione dell'incertezza e della instabilità. Allora archiviamo questa discussione e concentriamoci sul resto, a cominciare dai progetti sul *recovery fund*, con il pieno protagonismo del Parlamento e il coinvolgimento delle Regioni e delle Province autonome. Non escludiamo, inoltre, per puri motivi ideologici, la possibilità di ricorrere al MES sanitario. Nella bozza di piano le spese sanitarie sono al sesto posto, con un impegno di 9 miliardi, quando se ne vogliono destinare 74 alla transizione ecologica e 50 alla digitalizzazione e all'innovazione; molto bene, però sono appena 9 miliardi dopo tutto quanto è successo in questi mesi, che ci ha ricordato l'importanza di una sanità a 360 gradi, dalla medicina di base ai reparti avanzati, alla ricerca, alla necessità di garantire davvero su tutto il territorio nazionale livelli essenziali di assistenza. Facciamo una valutazione nel merito, in base alle reali esigenze dell'Italia; mettiamo da parte le questioni ideologiche, ragioniamo in maniera pragmatica. La pandemia ci ha insegnato soprattutto questo Signor Presidente, signor Presidente del Consiglio, onorevoli colleghi, noi oggi non votiamo solo la riforma del MES, ma decidiamo se siamo un Paese affidabile che dà seguito agli impegni assunti o se invece siamo solo dei parolai che non tengono fede alla parola data e mettono in discussione l'Europa; quell'Europa che ci sta aiutando a risolvere e a risollevarci dalla crisi da Covid e sta per metterci a disposizione la bellezza di 82 miliardi di euro a fondo perduto e 127 miliardi di euro in prestito. soldi veri, il valore di dieci manovre finanziarie che serviranno a tutelare posti di lavoro, a salvare aziende dal fallimento, a togliere famiglie dalla disperazione; soldi che noi chiediamo vengano spesi attraverso scelte oculate e trasparenti del Governo, su impulso e sotto il controllo del Parlamento, senza bisogno di doversi inventare fumose *task force,* né di doverne attribuire l'improbabile paternità all'Europa. È ora che prendiamo una decisione, anche perché abbiamo già tenuto bloccato il Paese e l'Europa sin troppo per mesi, sia sull'uso del MES sanitario, che sulla riforma del Meccanismo europeo di stabilità oggi all'ordine del giorno. Sono due questioni diverse, entrambe di grande rilievo, perché non si può continuare a ignorare la drammatica situazione sanitaria in cui ci troviamo e ad insistere nel porre veti per motivi puramente ideologici. Con diverse centinaia di morti al giorno per Covid è criminogeno ostinarsi a non voler ricorrere ai fondi del MES sanitario, perché ne va della vita di migliaia di persone *(Applausi)* e sarebbe autolesionista opporsi alla riforma del Meccanismo europeo di stabilità, che non è altro che uno strumento di finanziamento sulla cui modifica non dovrebbero esserci dubbi, dal momento che i cambiamenti apportati ne migliorano l'efficacia che abbiamo contribuito noi stessi come Paese a formularli. Ciò che viene introdotto rispetto all'eventuale ricorso al MES in caso di crisi bancarie serve all'Europa e può rivelarsi molto utile alla stessa Italia, perché l'onere di far fronte ad eventuali problemi finanziari delle banche non viene lasciato ai singoli Stati, ma viene coperto con risorse europee, cioè introduce un sostegno comune condiviso da tutti. Trovo piuttosto stucchevole la discussione se questa riforma serva di più all'Italia o ad un altro Paese. Questa riforma serve al sistema bancario europeo nella sua interezza, il il che è molto positivo, e se le banche italiane dovessero entrare in difficoltà, come di certo non ci auguriamo, con questo meccanismo avremmo una sorta di paracadute, a difesa del sistema finanziario dell'intero continente e di quello italiano. Per questo è populista continuare a rallentare un percorso che è utile agli italiani, oltre che agli europei tutti. Noi di Italia Viva non abbiamo dubbi: siamo a favore del Meccanismo europeo di stabilità e della sua riforma e troviamo logico che l'intera maggioranza riconfermi oggi l'identità europeista di questo Governo, votando a favore. Allo stesso modo riteniamo logico ed urgente ricorrere al MES sanitario, che ci aiuterebbe ad evitare enormi sofferenze ai singoli come al Paese. Il Consiglio europeo di domani è cruciale per una serie di ulteriori motivi, a partire dalle questioni legate alla politica estera. Innanzitutto, è necessario che l'Unione europea non si pieghi al *Diktat* di Polonia e Ungheria. Apprendiamo con piacere, signor Presidente, dal suo intervento che si starebbe per pervenire ad un accordo; la cosa sarebbe positiva, ma solo a patto che non si facciano concessioni sul mancato rispetto dello Stato di diritto. L'Italia deve dirlo chiaramente: i soldi per la ripresa post pandemia sono preziosi, ma non siamo disposti a farci ricattare pur di ottenerli attraverso il venir meno dei valori fondanti dell'Europa. L'Unione europea non deve fare sconti a nessuno rispetto alla tutela dei diritti. Pertanto, condividiamo il rinnovo delle sanzioni contro quei Paesi che continuano sistematicamente a violare i diritti umani, così come condividiamo il duro richiamo alla Turchia al rispetto del diritto internazionale. Grande attenzione va anche rivolta alla vicenda Brexit, come pure a tutte le questioni sulla sicurezza. Ricordo che il 14 dicembre ricorre l'anniversario della morte di Antonio Megalizzi, ucciso due anni fa, in un attentato terroristico a Strasburgo. In conclusione, signor Presidente, bisogna affermare un messaggio forte, positivo e rincuorante: l'Europa c'è, l'Europa oggi ci offre importanti opportunità e noi di Italia Viva chiediamo di avere il buon senso di usare queste opportunità per il bene degli italiani e delle prossime generazioni. *(Applausi).* presidente Conte ha un'alta considerazione di se stesso e nessuna considerazione del popolo italiano. Nel suo intervento e anche nella risoluzione di maggioranza vi è tutto e nulla, manca la verità e manca ogni visione, mentre oggi vi è disperato bisogno di verità e di visione. I suoi alleati dicono che abbia troppi poteri e forse ambisce ad avere tutti i poteri. Ha spazzato via la stampa e il ruolo dell'informazione con la diretta Facebook, come se l'Italia fosse un grande fratello; ha svuotato il Parlamento con DPCM, decreti a raffica e fiducie poste per coartare ogni dissenso. Sta cercando ora di esautorare il Governo con la cabina di regia sulle risorse del *recovery fund,* il tesoro che considera il suo tesoretto. In questo appare come Gollum nella saga «Il Signore degli Anelli»: il mio tesoretto. Aveva detto che glielo aveva chiesto l'Europa. Quest'ultima lo ha clamorosamente smentito. Presidente Conte, il partito dell'uno vale uno, il suo partito, ha di fatto consegnato tutto il potere ad uno, tutto a lei e ogni qualvolta vi sia da decidere una nomina, a sua volta, lei nomina una *task force* di tecnici che svuotano le Istituzioni; tecnici, alla faccia dell'uno vale uno e il suo partito la applaude come se fosse il suo fondamento. Oggi solo il MoVimento 5 Stelle lo ha applaudito durante il suo intervento. Gli altri esponenti della maggioranza sono stati fermi, salvo ovviamente nell'ultimo applauso, quello che non si nega a nessuno. Si chieda perché l'abbia applaudito Presidente Conte, lei ormai non ha limite nelle sue ambizioni e quindi le cito con rispetto quello che lei pensa essere stato un suo collega, magari, minore, sicuramente, ai suoi occhi, minore. Abraham Lincoln nel 1858 affermava: «Potete ingannare tutti per qualche tempo e qualcuno per sempre, ma non potete ingannare tutti per sempre». Mi rivolgo ora al suo partito, ai senatori del MoVimento 5 Stelle citando un successore più recente di Lincoln, John Kennedy, che riportando proprio quella celebre frase di Lincoln, aggiunse, come se parlasse a quest'Assemblea, a voi del MoVimento 5 Stelle, «il massimo della stupidità si raggiunge non tanto ingannando gli altri, ma ingannando se stessi, sapendolo». Ebbene, qui si inganna e voi vi ingannate, ben sapendo di mentire a voi stessi. Il Governo ha mentito un anno fa al Parlamento, quando affermò che nulla era ancora deciso e che vi erano margini per trattare. Così non era e così non è stato, perché non vi è nulla di nuovo e significativo rispetto a quanto tutti sapevamo un anno fa. Il presidente Monti ha definito questo passaggio

Tutto era quindi già deciso nel novembre del 2019. Era però falso che fosse a beneficio del Paese. Tanto è vero questo, che persino lei afferma e i suoi sostenitori giurano - dovremmo dire spergiurano - che mai l'Italia ne farà uso. Se è a nostro beneficio, perché mai non dovremmo utilizzarlo o escludere di farlo?

Presidente, il suo secondo Governo nacque su questo, su una grande menzogna, e cerca di sopravvivere oggi con un'altra grande menzogna.

Questo fatto, signor Presidente, mina il rapporto di leale collaborazione che dovrebbe essere a fondamento del confronto tra Governo e Parlamento. Il partito di maggioranza relativa del suo Governo dice inoltre che non attiverete nemmeno la linea sanitaria. In realtà, avete già deciso di attivarla, ma non lo comunicate nemmeno oggi, anzi, lo negate. Ancora una volta, negate e celate la realtà anzitutto a voi stessi e vi ingannate. Avete già

Speranza vi aveva chiesto 58 miliardi e voi ne date 9. Come mai non li avete previsti? Perché avete già deciso di utilizzare a questo scopo proprio la linea sanitaria del MES. Lo avete già deciso, ma lo nascondete ancora oggi al Parlamento e lo celate al Paese. In fatto di bugie siete campioni: siete la coalizione e il Governo di Pinocchio, il gatto e la volpe. La storia ci dirà chi è il gatto e chi la volpe e dove sono finiti i trenta denari. Nel merito, il MES ha tre aspetti. Vi è anzitutto il salva Stati, con degli Stati che sono più uguali degli altri. Altro che uno vale uno! Vi sono alcuni Stati che vi possono ricorrere senza pagare pegno (i loro Stati) e gli altri che, se vi ricorrono, vengono commissariati (noi). il salva banche, con delle banche più uguali delle altre (quelle dei Paesi in regola con i vincoli europei, cioè i loro Paesi e le loro banche). È facile intuire a cosa serva ed è facile capire che la riforma del MES, con questa nuova strumentazione, debba essere varata prima della Brexit, perché non si sa mai cosa possa accadere a quel punto. Il salva banche non vi era durante la crisi greca,

con macelleria sociale che non ha pari e con misure imposte dai banchieri per salvare i loro forzieri che nemmeno un Governo di occupazione avrebbe mai osato fare; tutto per garantire il salvataggio delle banche francesi e tedesche e i loro profitti. Sulla base di quell'esperienza drammatica ora si sono fatti più furbi, anche perché lo strumento è talmente squalificato che nessuno si azzarda a sollecitarlo. Parlano - e non a caso - di stigmate greche, evocando quindi le ferite comparse sul corpo di Cristo, per far capire di cosa si parli e quanto sia inviso lo strumento. Il fine è però sempre lo stesso: salvare le banche tedesche e francesi, ove ve ne fosse bisogno. Questa riforma serve a loro, che hanno nella loro pancia montagne di derivati. Sapete che solo Deutsche Bank possiede 50.000 miliardi di euro di derivati? Se mai dovesse scoppiare la bolla, travolgerebbe il sistema finanziario tedesco. Il terzo aspetto è il MES sanitario. Non fa parte della riforma, ma la accompagna. Anche qui avete mentito. Il MES sanitario in cinque mesi, malgrado la pandemia, nessun Governo si è sognato...

del suo debito e della sua mancata crescita, di cui siete responsabili, potrebbe essere costretta ad attivarlo. L'Italia non è certamente Siamo molto più appetibili: non abbiamo solo porti e aeroporti, che Cina e Germania si sono già spartiti in Grecia; abbiamo la cassaforte del risparmio europeo, che fa gola a molti; abbiamo un sistema agricolo, agroalimentare e industriale che fa gola soprattutto oltralpe. Voi state creando tutte le premesse, con un incontrollabile debito pubblico, e tutte le condizioni giuridiche, anche con questa riforma del MES, per farci fare la stessa sorte della Grecia, ovviamente con strumenti e metodi diversi, ma simili negli effetti...

Signor Presidente, signor Presidente del Consiglio, onorevoli colleghi, la riunione del Consiglio europeo prevista per il 10 e 11 dicembre affronterà il tema delle risposte europee alla pandemia e vedrà i capi di Stato e di Governo chiamati a occuparsi di un'agenda impegnativa e complessa, che va dai cambiamenti climatici alla sicurezza, alla lotta al terrorismo, alle relazioni dell'Unione europea con la Turchia e con il Sud del Mediterraneo, per concludersi con il vertice euro dedicato all'unione bancaria e all'unione dei mercati di capitali esteso ai 27 Paesi. Il prossimo vertice avrà all'ordine del giorno anche la riforma del trattato MES. Così come approvata nell'ultima riunione dell'Eurogruppo, la riforma a mio avviso, ha ancora alcuni punti deboli. Pur condividendo la parte relativa all'introduzione anticipata al 2022 del sostegno comune al Fondo di risoluzione unico per le banche, sinteticamente detto *common backstop*, ritengo più complessa, invece, la vicenda che riguarda le modifiche delle clausole di azione collettiva e la revisione delle linee di credito, su cui ci sono ancora dubbi da risolvere. Così come approvate in Eurogruppo, queste modifiche sono negative per il nostro Paese, soprattutto quelle riguardanti i requisiti di accesso al MES, come la reintroduzione dei parametri di stabilità e crescita e il *fiscal compact*. Approvando la riforma, così com'è scritta, si accetterebbe la configurazione del MES come strumento che interviene solo a favore degli Stati che di fatto non ne hanno bisogno, penalizzando Paesi come l'Italia, con un debito elevato. Oggi, dopo aver archiviato una fase negoziale lunga e difficile, è fondamentale che le risorse finanziarie a sostegno dei piani nazionali di ripresa affluiscano secondo la tempistica prospettata, alla quale i Paesi membri hanno affidato in larghissima parte le aspettative di ripresa economica. Parliamo di 209 miliardi di risorse, che sono un'enormità, un ordine di grandezza senza precedenti e una grandissima opportunità, che non dovrebbe consentire margini di errore, ritardi o dispersioni. Il Parlamento e il Governo sono responsabili di queste scelte e ne rispondono al Paese e al popolo. Non esito a definire epocale il voto al quale siamo chiamati oggi. Abbiamo conosciuto bene la vecchia Europa, quella della *troika*, del programma micidiale che ha messo in ginocchio un Paese come la Grecia. All'indomani della crisi del 2007-2008 l'unico modo che l'Unione europea ha trovato per reagire è stato un'iniezione massiccia di austerità, che dobbiamo superare. Per correggere quella filosofia, il programma del Movimento 5 Stelle, all'epoca in cui siamo stati candidati, si impegnò a modificare radicalmente queste istituzioni. Attualmente il MES non è, come si vorrebbe far credere, un'istituzione che fa capo direttamente all'Unione europea, bensì un meccanismo intergovernativo e non elettivo, che ha un enorme potere di influenza nelle scelte nazionali, senza avere tuttavia una legittimazione politica. Nessun Paese sinora vi ha fatto accesso. In tanti ritengono che l'attivazione in ambito sanitario...

in questa situazione di tranquillità la BCE ci potrà aiutare, ma non dimentichiamo che in questo triennio il Governo ha previsto che il nostro debito pubblico aumenterà di circa 500 miliardi e la velocità di crescita del debito sarà superiore a quella di crescita del PIL. che, se attivassimo oggi linee di credito legate al MES, ci sarebbero condizionalità molto lesive per l'Italia. Riteniamo che il Governo si stia muovendo adeguatamente, perché l'Europa di domani deve essere inclusiva, solidale, rispettosa della sovranità e sostenibile, senza istituzioni non elette che monitorano, controllano e di fatto impongono la loro visione globalizzata e ultraliberista. Per questo motivo, ho sottoscritto la proposta di risoluzione n. 6, che vincola in maniera assoluta l'introduzione di modifiche all'attuale testo, nella direzione di valutare i prerequisiti dell'accesso alle linee di credito, escludendo in maniera chiara ogni meccanismo automatico di ristrutturazione dei debiti. *(Applausi)*. PRESIDENTE.

Mi riferisco al nostro rapporto con l'Unione europea. Poco più di un anno fa, l'Italia si trovava a camminare lungo il viale di un pericoloso isolamento, grazie a chi invocava pieni poteri dalle spiagge del Papeete e strizzava l'occhio a Orban e al restante gruppo di Visegrád. Si trattava, è bene ricordarlo, di un vero e proprio tradimento della tradizione europeista, di cui la nostra Repubblica è fedele baluardo, tradimento al quale abbiamo reagito. È proprio questo, se vogliamo, che segna un solco profondo di discontinuità tra l'Esecutivo attuale e quello precedente. Da una parte, infatti, troviamo chi - oggi per fortuna non più al Governo del Paese - fa il tifo per le democrature e, dall'altra, chi invece difende la democrazia e lo Stato di diritto.

certo non possiamo nascondere quanto acceso e critico sia stato il dibattito degli ultimi anni sul tema europeo, sul rapporto da tenere con l'Unione, sull'identità dell'istituzione e sulle sue relazioni con i Paesi membri (un rapporto piuttosto contrastato, soprattutto a causa di alcune politiche economiche della zona euro). Alcune questioni le abbiamo poste anche noi come Paese Italia: lo abbiamo fatto con forza, liberando il dibattito dalla domanda se occorra stare dentro o fuori dall'Europa, interrogandoci però su come cambiarla e migliorarla. infatti tutti consapevoli che la costruzione europea necessiti di un generale ammodernamento, ma anche che i progressi maggiori si sono sempre registrati durante i periodi di crisi. Ne abbiamo avuto ulteriore prova anche in questo tormentato 2020, in cui la pandemia da Covid ci ha messo in serie difficoltà. Consentitemi per un attimo, però, di tornare alle politiche dell'Europa e alle evoluzioni avvenute. Si è dibattuto a lungo sul fatto che le regole di bilancio fossero troppo stringenti e il Patto di stabilità e crescita è stato sospeso. Si è ritenuto che le regole sugli aiuti di Stato fossero troppo rigide e sono state sospese. Si è lamentato che la BCE fosse troppo attenta al lato dell'inflazione e oggi abbiamo il Pandemic emergency purchase programme Si è ventilata infine la necessità di dotare l'Unione europea di emissioni comuni e abbiamo ottenuto il meccanismo Sure e il *recovery fund*. Mi vengono in mente questi quattro aspetti per affermare i passi in avanti compiuti lungo il percorso di una nuova costruzione europea; sono punti e aspetti che certamente non possono restare temporanei e che andranno consolidati anche dopo la fine della pandemia, ma che sarebbe un errore non riconoscere. Dico di più: se volessimo con onestà intellettuale richiamare l'enorme portata della risposta europea alla crisi pandemica, che è anche un manifesto politico, ci basterebbe richiamare il Next generation EU. Abbiamo infatti invocato per tanto tempo gli eurobond e ora abbiamo *bond* europei per realizzare politiche finalmente espansive, una risposta politicamente robusta, che non dobbiamo sprecare e che obbliga a un impegno diretto le principali istituzioni democratiche. Ecco perché qui in Senato ci siamo assunti da subito la responsabilità di sottolineare la centralità del ruolo del Parlamento, chiedendo con forza di sottrarre le linee guida del piano all'idea di comprimerle a semplice allegato alla NADEF, dando corso a un lavoro a tamburo battente condotto dagli organismi parlamentari che ha restituito al Governo un documento qualificato, poi consegnato e apprezzato in Europa. Allo stesso modo, oggi torniamo a chiedere che la discussione sull'impianto di investimenti e riforme e sulla *governance* resti di assoluta centralità, perché non è pensabile procedere senza un reale coinvolgimento dell'organo che è espressione per eccellenza della rappresentanza democratica. Non è solo logico, ma è giusto che ai parlamentari eletti venga riconosciuto venga riconosciuto a pieno titolo di essere parte attiva nelle scelte che dobbiamo assumere per il futuro. Il perché di questa richiesta non è quindi un vezzo o un capriccio, né tantomeno può essere additata come un'iniziativa che vuole mettere in discussione la necessità di proseguire sulla strada tracciata con questo Governo e con questa maggioranza. Significa semmai voler rafforzare l'azione di un Governo, il nostro, nato su iniziativa parlamentare e che ha la necessità di continuare a condividere con il Parlamento obiettivi e metodi di lavoro, ma anche strumenti per poter vincere la sfida che abbiamo davanti

Stiamo spendendo oggi i soldi dei nostri figli e dei nostri nipoti, proprio per lasciare loro un'organizzazione dello spazio pubblico più verde, più resiliente, più inclusiva e più giusta. Non possiamo consegnare i processi selettivi e decisionali a visioni squisitamente tecnocratiche, ma dobbiamo liberarli a una discussione vera e politica dell'idea di Paese che vogliamo ricostruire. Farlo anche qui, in Parlamento, significa farlo meglio, assicurando il contributo di chi caparbiamente continua a lavorare su orizzonti di inclusione e di sviluppo, lì dove il sovranismo, invece,

sessione del 10 e 11 dicembre, tratterà tanti temi e tanti temi importanti per il futuro dell'Europa: il Meccanismo europeo di stabilità, con la modifica del Trattato, grandi questioni di politica estera, il Covid-19, la sanità e i vaccini, il clima. Il dibattito nazionale non ha avuto particolare enfasi né su estero, né su clima, né su pandemia. estero è molto importante: vorrei ricordare che riguarda i rapporti con la Cina e con gli Stati Uniti, l'espansionismo della Turchia, la questione del Mediterraneo connessa a immigrazione, terrorismo e anche approvvigionamento energetico per il nostro Paese. il clima, con gli obiettivi del 2030, i vaccini e le restrizioni, che creano un po' di confusione nel nostro Paese. Si è discusso solo di MES e neanche di Trattato;

per non chiederlo», per mantenere ancora questo Governo che non lo chiede. Noi, invece, interveniamo nel dibattito per discutere il merito, che è il Trattato. Dopo il 2012 è stato chiaro a

Nel 2017, infatti, si è iniziato un percorso di modifica, con il dibattito sul modello intergovernativo o comunitario; prevalse il primo. Nel 2019, il preaccordo non è stato soddisfacente. Il nostro presidente Il nostro presidente Silvio Berlusconi, nel dicembre 2019, denunciava il nostro dissenso e chiedeva una riforma complessiva che portasse trasparenza e democrazia nei processi decisionali. Perché critichiamo?

Se a qualcuno sembra possibile, lo dica. Per l'altra linea di prestito, la condizionalità rafforzata, legata a un programma di riforme che comprende la ristrutturazione del debito, con la rimodulazione coatta delle sue scadenze o la diminuzione del valore nominale, che fine farebbero i risparmi delle famiglie italiane?

clausole di azione collettiva, a votazioni singole o per numero o per quote: l'Italia può andare in minoranza con il voto di Stati che valgono singolarmente un suo ventesimo? Noi, Noi, uno dei quattro grandi, tra i fondatori! Può andare in minoranza, tolto il caso dell'emergenza, perché ha il 17,70 e quindi non supera il 20 Questo è l'altro quesito che pongo, sulla *governance*: totale emarginazione della sfera politica dal processo decisionale (ho apprezzato l'intervento del collega Stefano, che è della maggioranza) con potere di immunità per il direttore generale; questo, aggiunto al sistema di voto, porta L'Italia a non essere determinante e non lo sono nemmeno il Parlamento europeo e la Commissione.

Signor Presidente, colleghe e colleghi, noi crediamo nell'Unione europea, che in fondo è il frutto di quella Comunità economica per il carbone e l'acciaio, poi CEE, nata a Roma nel 1958, che ha dato unità all'Europa e bene comune. Noi vogliamo il MES, vogliamo il MES riformato. Non sfugge però a nessuno che, come per la Grecia, con il Covid-19 si è sospeso il meccanismo del MES, MES, come pure quel meccanismo che adesso viene riproposto, perché non funziona tecnicamente, perché è ancorato al Fiscal Compact, non praticabile per tutta l'Europa. Crediamo nell'Unione europea che ha avuto la capacità, con la pandemia, di fare un salto di qualità, un debito comune, i cosiddetti eurobond, che richiamano Giulio Tremonti, Ministro del Governo Berlusconi dieci anni orsono. Questo è il solco, il vero passaggio federale contro gli egoismi dei Governi e della burocrazia. Che senso ha sottoscrivere un Trattato sapendo fin d'ora che non lo si potrà rispettare? È come sposarsi per provare se funziona il divorzio, Noi, Paese fondatore, dobbiamo andare oltre. Il *recovery fund* dimostra che si può e anche il MES per la sanità dimostra che si può, perché fu in deroga al primo MES. Qualcuno dice che prevale la questione politica. Noi facciamo prevalere, in questo caso, la questione di merito su quella politica: siamo contro il suo Governo, non dobbiamo ripeterlo. Diciamo però che il Governo non ha trattato e, preso dalle liti interne dei commissari, non concretizza nulla sul *recovery fund*, galleggia e non viaggia, si può dire, perché effettivamente è questo lo stato. In conclusione, onorevoli colleghi, ci rendiamo conto che in una trattativa complessa non tutto è possibile, ma non dobbiamo rinunciare agli interessi nazionali. Accontentarci con il detto «piuttosto che niente, meglio piuttosto» non va bene, non va assolutamente bene. *(Applausi)*.

Signor Presidente, breve riassunto delle puntate precedenti: 19 luglio 2012: seduta n. 669 della Camera - ratifica ed esecuzione del *fiscal compact* - onorevole Giorgetti in dichiarazione di voto finale: «La parte politica che le parla in questo momento è a favore dell'Europa (...) ma voterà contro il *fiscal compact*. (...) Senza crescita economica un debito pubblico come quello italiano non è sostenibile. Non si tratta soltanto della speculazione internazionale, ma semplicemente della naturale osservazione che, non crescendo e non producendo ricchezza, nessun debito può essere rimborsato». 2.889 giorni dopo, il 16 giugno 2020, il professor Romano Prodi in audizione presso la XIV Commissione della Camera: «Finalmente si corregge l'errore tragico che ha reso molto più grave del dovuto la scorsa crisi, che ha danneggiato fortissimamente l'Italia e che ha addirittura sfasciato l'economia greca. Parlo dell'austerità».

«Il *fiscal compact* va nella giusta direzione, ma lo hanno approvato solo oggi; poi ci sarà il rinvio e si rischia di avere un patto che avrà meno impatto di quello prospettato». Nel 2012 al PD l'austerità andava bene, anzi l'avrebbe voluta prima; solo la Lega era contraria. Oggi sono tutti i contrari. *(Applausi)*. A differenza dell'Europa, che ha molti padri, l'austerità ora non ne ha nessuno.

Un uomo brioso come la sua punteggiatura. *(Applausi).* Pochi secondi dopo, onorevole Borghi: «Questa la salviamo da dare ai risparmiatori della prima banca che salterà. Tiferò per gli inseguitori». È ancora su Twitter, andatela a vedere. 685 giorni dopo, il 4 novembre 2015, nella 6a Commissione parere al decreto legislativo di recepimento del *bail in*, il resoconto sommario riporta che il senatore Tosato rimarca «i rischi cui potranno essere esposti risparmiatori e, in particolare, i correntisti, senza che tale intervento sia peraltro risolutivo delle crisi bancarie». giorni dopo fu pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* il decreto-legge salva banche (non devo dirvi che cos'è). Sei giorni dopo, il 28 novembre 2015, a Civitavecchia si tolse la vita Luigino D'Angelo, obbligazionista di Banca Etruria, ex dipendente dell'Enel, per anni iscritto alla CGIL. La moglie ricordò che era sempre stato un uomo di sinistra. 914 giorni dopo, il 30 maggio 2018, nella dichiarazione dell'Autorità bancaria europea sul trattamento degli strumenti finanziari soggetti a *bail in* venduti a piccoli risparmiatori (cioè il caso del povero Luigino D'Angelo), «anche in assenza di *miss-selling*, le conseguenze dell'applicazione del *bail in* ad obbligazioni subordinate, in caso di esposizioni significative, potrebbero presentare delle sfide specifiche dal punto di vista degli effetti di contagio e della stabilità finanziaria». maggio 2018 disse che il *bail in* destabilizzante era stato un errore. Ovviamente, col semaforo verde dell'Europa, arriva, come al solito dopo, il PD. Il 9 Aprile 2019, Vincenzo Visco, in un'intervista a «LaVerità» stato «un grave errore di Letta accettare il *bail in* retroattivo delle banche. Capisco che c'erano pressioni, si è parlato addirittura di ricatto, tuttavia bisognava dire di no a Wolfgang Schäuble». Quindi, ricapitolando, per il PD e per Bankitalia l'unione bancaria era una buona cosa. Per cambiare idea, il PD ha aspettato che fosse l'Autorità bancaria europea a dire che i risparmiatori italiani erano stati usati come cavie.

«Oggi state commettendo un grave errore sottovalutando la portata di questo provvedimento. Queste sono decisioni che condizioneranno per sempre la nostra vita e quella dei nostri figli; decisioni che cambieranno la nostra autonomia in sede economica, di bilancio e fiscale». Queste parole le teniamo così come sono: si applicano perfettamente all'oggi, ancora di più per i motivi dettagliati dall'onorevole Borghi alla Camera. Mi avvio a concludere. Rinuncio a rivolgermi al partito di maggioranza relativa, per il semplice motivo che oggi ha perso agibilità politica. I traditori fanno comodo a qualcuno, ma tutti ne diffidano, e quindi *de hoc satis*. Parliamo invece al PD, l'unico pezzo dell'attuale maggioranza che un futuro politico ce l'avrà e col quale quindi è necessario dialogare. Dopo l'austerità, dopo il *bail in*, anche con la riforma del MES (che è l'austerità), andrà a finire come diciamo noi. E anche questa volta voi andate dritti per la vostra strada. Forse vi stanno ricattando oppure, più semplicemente, pensate che toccherà a noi macellare i risparmiatori. Ma lo pensavate anche al tempo del *bail in*, e invece il sangue dei risparmiatori italiani è sulle vostre mani e ci avete anche perso le elezioni. Quindi, non ci aspettiamo di convincervi, non ci interessa. Ma c'è una cosa che deve interessare voi: che cosa hanno in comune il *fiscal compact* e il *bail in*, i due errori che avete già ammesso? È molto semplice: sono due parolette in inglese di cui l'opinione pubblica si disinteressava, perfino io, che sono del mestiere e che dal giugno 2013 mettevo in guardia contro i pericoli del *bail in*, ignoravo la discussione che si stava svolgendo in Parlamento e le parole lungimiranti dei colleghi Giorgetti, Bitonci e Tosato, ma potrei aggiungere Garavaglia e tanti altri. Da allora qualcosa è cambiato, e concludo: da allora, purtroppo per voi, cari amici del PD, c'è stato un dibattito nel Paese. Il livello di consapevolezza dell'elettorato non è più quello del 2012, quindi oggi migliaia di occhi ansiosi guardano a questa discussione con attenzione e aspettano l'esito del voto per dividere questo Parlamento in due categorie: i patrioti e i traditori *(Applausi)*. Nonostante tutti gli sforzi dell'antipolitica per confondere le acque e offuscare le responsabilità, oggi sarà chiaro chi è dalla parte della libertà e del Paese e chi è dall'altra parte. Vi faccio i miei auguri.

onorevoli cittadini che ci ascoltate da fuori. Vede, presidente Alberti Casellati, faccio questo appello anche ai cittadini perché in questo periodo di Covid - sono sincero - la presenza in Aula degli ospiti, che prendevano

È stata una discussione molto lunga e anche partecipata (solitamente la discussione generale non è un momento troppo partecipato). Ho ascoltato tutti gli interventi dei colleghi, anche quelli di opposizione.

partendo dall'ultimo, quello del senatore Bagnai, del quale spesso ho apprezzato alcuni passaggi, non sicuramente la parte finale - ci sono stati aspetti condivisibili. Poi, c'è stato il senatore Candiani, che personalmente mi fa molta simpatia,

Via i cartelli!

ringrazio, signor Presidente, le chiedo solo gentilmente di recuperare questi due minuti di interruzione. Stavo dicendo, a proposito del senatore Monti, che, durante il suo intervento, ha fatto riferimento ai parlamentari del MoVimento 5 Stelle e sedendo tra i senatori del MoVimento 5 Stelle, si è fatto l'impressione che il MES non sia un argomento impossibile, ma che ci sia era bisogno di un impegno di pedagogia didattica. *(Applausi)*. Vede, presidente Monti,

sta facendo con lei: il prossimo passo sarà quello di votare con noi un bel no al MES, e il suo percorso di ripetizioni sarà concluso.

oggi non si vota il MES. Questa è la prima cosa da mettere a parte. Noi riteniamo, come MoVimento 5 Stelle, che questo sia uno strumento veramente d'altri tempi, uno strumento anacronistico. È uno strumento che non serve. Purtroppo

nel loro partito ci sono i padri e le madri del MES, perché nel 2011 in Europa andarono loro a votarlo e non il MoVimento 5 Stelle *(Applausi)*. Su questo siamo d'accordo, colleghi, anche con l'opposizione. Poi ci sta anche parte della maggioranza che legittimamente è convinta che questo strumento possa essere utile, così come più volte tutti abbiamo detto. Al momento opportuno il Parlamento sovrano si esprimerà

europea; noi siamo più per una comunità che sia più vicina ai cittadini. In questo periodo difficile di Covid finalmente si è trovata quella chiave che era mancata in tutti gli anni precedenti e che ci consentirà di avere un'Europa dei popoli, un'Europa che sia realmente vicina ai cittadini. *(Applausi)*. Noi crediamo che questo percorso sia possibile anche con le diversità che in questo momento sono all'interno Se oggi dovessi dare un titolo al mio intervento, lo chiamerei «voce di popolo», e non perché mi senta portavoce del popolo; nei Palazzi si chiamano «voci di corridoio» e nei giornali si chiamano *rumors*. Conte, un fatto che la riguarda e che qualche giorno fa mi è capitato. Un mio amico ha una piccola azienda ittica: esce il pomeriggio con la barca, cala le reti e la mattina successiva porta il pescato in porto; è uno di quei cittadini italiani

(Digli a Conte di andare avanti e non voltarsi indietro, perché dietro il popolo ha capito il prezioso lavoro che lei sta facendo). *(Applausi)*. Quindi, a lei, presidente Conte,

Signor Presidente, mi accingo a completare il mio intervento. Lo dico anche per i nostri detrattori: è vero che sul MES il MoVimento 5 Stelle ha avuto un momento di estrema difficoltà. Lo sappiamo, è difficile. Compagni del MoVimento 5 Stelle, compagni di squadra del MoVimento 5 Stelle, credo sia arrivato il momento di prenderci per mano. Anzi, prendiamoci per gomito, perché per mano non possiamo, e andiamo avanti e non fermiamoci. Concludendo, signor Presidente, in questi giorni mi riecheggia nella mente un'immagine. Ricordo il grande Dario Fo

«Fatelo voi, per favore. Fatelo voi!» Lo dico al MoVimento 5 Stelle: è il momento di continuare e non di dividerci.

Avverto che sono state presentate le proposte di risoluzione n. 1 (testo 2), dai senatori Licheri, Marcucci, De Petris, Unterberger e Faraone, n. 2, dalla senatrice Bonino e da altri senatori,

Signor Presidente, colleghe e colleghi, membri del Governo, presidente Conte, l'Italia è la principale beneficiaria di uno straordinario atto di solidarietà dell'Europa. E' la stessa Italia dovrebbe bloccare la riforma di uno strumento, su cui sono d'accordo tutti gli altri Paesi e tutte le principali famiglie politiche europee, una riforma che protegge le banche, richiesta proprio dagli Stati del Sud Europa e più volte adeguata alle esigenze italiane? Tutto questo con argomenti assurdi, come quello secondo cui, con la riforma, verrebbero presi i soldi italiani per aiutare le banche tedesche. Come ricorda Cottarelli, casomai è lo Stato italiano e non quello tedesco ad avere bisogno di aiuto in caso di crisi delle proprie banche. Inoltre, questi sono gli stessi argomenti che hanno usato i cosiddetti Paesi frugali contro gli aiuti all'Italia, dal loro punto di vista eccessivi. Come spiego alla parrucchiera che deve pagare con le sue imposte i debiti degli italiani? Questo aveva ripetuto più volte il cancelliere Kurz quando si trattava sul *recovery fund.* Adesso questa argomentazione nociva per la solidarietà europea la vogliamo usare proprio noi che in questo momento abbiamo più bisogno dell'Europa? Vogliamo legittimare il veto di Polonia e Ungheria sul *recovery fund,* ponendo anche noi un veto in un altro campo? Sono contenta che si sia trovata una mediazione almeno nella maggioranza. Bloccare l'intera eurozona su modifiche marginali di un trattato avrebbe avuto davvero dell'incredibile, per non parlare della confusione di questo dibattito partiti che non vogliono né la linea del MES sanitario, né la riforma del MES; altri che vogliono sia la linea sanitaria del MES sia la riforma del MES; partiti che sono favorevoli al MES sanitario, ma sono contrari alla riforma del MES; partiti che accettano la riforma del MES, ma non vogliono attivare quello sanitario. Tutto questo è già difficile da spiegare agli italiani: immaginate come viene visto negli altri Paesi. Lì nessuno discute del MES e il dibattito italiano viene raccontato con termini come commedia, psicodramma, Paese che gioca col fuoco. Purtroppo, questo danno alla reputazione è la conseguenza della battaglia degli antieuropeisti che sognano di portare indietro le lancette del tempo, perché prima del Covid l'Europa era un bersaglio facile in grado di ingrossare facilmente il consenso a favore delle forze populiste. Covid, però, ha dimostrato che con gli egoismi e coi sovranismi non si salva nessuno e la logica del salvare gli altri coi propri soldi deve essere sostituita con la logica del salvare gli altri per salvare sé stessi. Questa è l'idea di fondo del MES, che con la riforma viene esteso anche al salvataggio delle banche in crisi. Che ci siano delle condizionalità va da sé, perché è legittimo che chi usa soldi propri per salvare altri possa porre anche delle condizioni. Ogni debito crea delle condizioni, come dice giustamente Giovanni Toti. Se ci battiamo per un cosiddetto nuovo MES, forse la cosa più importante sarebbe cambiarne il nome, perché ho la sensazione che alcuni non riescano più a liberarsi dai fantasmi che hanno creato con questo mostro propagandistico. In realtà, ci si salva solo con la solidarietà e con una sempre maggiore integrazione tra gli Stati membri, perché solo un continente di quasi 500 milioni di persone ha la forza economica e morale per affrontare una pandemia come quella che stiamo vivendo. L'Italia ha rischiato di assestare un brutto colpo al nuovo processo di integrazione e di mettere acqua nel mulino di quelli che parlano da sempre della sua scarsa affidabilità; un danno grande alla percezione dell'Italia sia sotto il profilo dell'affidabilità e istituzionale che dei suoi conti pubblici. Non ci poteva essere *spot* peggiore; non ci poteva essere regalo migliore a chi spera di poter tornare ai vincoli di stabilità e alla stagione del rigore finanziario. Sarebbe stato un gravissimo errore che, per fortuna, è stato evitato. Per questo il Gruppo per le Autonomie voterà con convinzione la proposta di risoluzione

le augurano buon lavoro e la invitano a schierare l'Italia dalla parte dell'europeismo, e non del sovranismo, nella importante discussione di giovedì e venerdì a Bruxelles. Davanti alla crisi pandemica l'Europa stavolta ha risposto battendo un segno positivo e il nostro Paese è protagonista di questa svolta. La riforma del MES è un piccolo passo in avanti, e va nella giusta direzione. Tuttavia, noi vogliamo prendere l'occasione di questo dibattito, al quale lei più volte ci ha richiamato, per utilizzare parole di verità e trasparenza - le stesse che ci diciamo negli incontri privati e in quelli di maggioranza - anche qui in Parlamento,

Certo, i problemi sono enormi (la distribuzione dei vaccini, il rapporto Stato-Regioni, i ritardi in tanti momenti importanti della vita del Paese), ma siamo per la prima volta a presiedere il G20. Come dice il nome, ricapiterà tra venti anni. E presiediamo il G20 nel momento in cui l'Italia può dettare la linea sul futuro economico post pandemia. Presiediamo il G20 nel momento in cui gli Stati Uniti tornano al multilateralismo; «*America* *is back*» è il titolo della politica estera di Joe Biden, il Presidente eletto.

Come non pensare che finalmente possiamo trasformare l'ambiente da mera questione, importantissima e ideale, a occasione di creare posti di lavoro, pensando che abbiamo con ENI, Enel, Snam, Saipem, le eccellenze della transizione energetica a livello non nazionale, ma mondiale. Quanti argomenti di discussione importanti. E lei, Presidente, li ha toccati. In questo i 200 miliardi del Next generation EU sono una grande conquista, ma sono una gigantesca responsabilità. allora essere chiari sul punto, e lo diciamo per il tramite del presidente del Senato al Presidente del Consiglio e a chi continua a sostenere che la posizione di Italia Viva sia legata a un qualche interesse di partecipazione alla cabina di regia. Noi non scambieremo il nostro sì alla proposta di *governance* in cambio di uno strapuntino o di un "aggiungi un posto a tavola". Detta in un altro modo, non già al Presidente del Consiglio che ne è consapevole, ma a chi ci segue, noi non stiamo minimamente chiedendo che nella cabina di regia ci sia anche un Ministro di un colore politico più vicino al nostro e lo dimostriamo in modo molto semplice. Ricordiamo agli

Avevamo detto che, di fronte ai 200 miliardi da spendere - cifra che non ricapiterà per anni, vorrei dire per decenni purtroppo o il Parlamento fa un dibattito vero, sfidando le opposizioni, oppure perdiamo la dignità delle istituzioni. C'è chi dice: «Ma come: durante la pandemia volete parlare di politica?». Eh già: già: se non parliamo di politica durante la pandemia, cosa ci stiamo a fare in Parlamento? *(Applausi).* Se davanti alla principale occasione per il futuro dei nostri figli non facciamo un dibattito parlamentare, con che faccia andiamo a sfidare le opposizioni?

Quello che non va bene, signor Presidente del Consiglio - e glielo diciamo guardandola negli occhi e in faccia - è che ci arrivi nottetempo, alle due, sulla posta certificata dei Ministri, un progetto di 128 pagine, che deve diventare un emendamento alla legge di bilancio, con una proposta che prevede dei *manager* con poteri sostitutivi rispetto al Governo e senza una discussione parlamentare, perché anche quest'anno la legge di bilancio non verrà discussa almeno da un ramo del Parlamento. Colleghi del Partito Democratico, eravamo insieme, nello stesso partito, quando due anni fa il presidente Conte e il vice presidente Salvini, uno di voi, uno di noi, attuale presidente *pro tempore* della Commissione affari costituzionali, addirittura firmò un ricorso alla Corte costituzionale contro la scelta del Governo di non farci discutere la legge di bilancio. Ora, tra quindici giorni accade la stessa cosa. Se una cosa la fa Salvini è sbagliata - non sempre, spesso, ma questo è un altro discorso - ma, se la facciamo noi, ed è la stessa, è ugualmente Non possiamo immaginare che, di fronte a una legge di bilancio non discussa, ci inseriamo, saltando e bypassando il Parlamento, tutta la principale discussione sul prossimo utilizzo

Signor Presidente, colleghi, 300 consulenti, quando si tagliano 300 parlamentari, sono la dimostrazione che si ha un'idea della politica che io non condivido.

Ritengo che un Governo non possa essere sostituito da una *task force.* Ritengo che un Parlamento non possa essere sostituito da una diretta Facebook. Ritengo che questa sia la battaglia di dignità che il Parlamento deve fare. Se questo è il Piano Marshall del futuro, dove sono i sindaci? Se questo è il Piano Marshall del futuro, dove sono gli esponenti del terzo settore? Se questo è il Piano Marshall del futuro non avrei mai immaginato di dirlo - dove sono le categorie e i sindacati? Non è immaginabile che, di fronte a 200 miliardi di euro, che vuol dire debito pubblico, noi rinunciamo a essere parlamentari. È chiaro questo? *(Applausi)*. Dopodiché, signor Presidente, parliamoci con chiarezza. È un problema solo di metodo? Magari. C'è qualcuno che, probabilmente, immagina che si possa "dipiciemmizzare" la politica. Ma c'è anche un problema di merito. Ho letto le carte del Next generation EU. Ma chi ha deciso che noi mettiamo nove miliardi di euro sulla sanità? euro sulla sanità? Questo è un passaggio importante. Giochiamo in maniera trasparente tra di noi. Quando il mio Governo, per tre anni, ha messo sette miliardi in più sulla sanità, tutti hanno detto, negli ultimi dieci mesi di *talk show*, che noi avevamo tagliato sulla sanità. In due anni e mezzo abbiamo messo più sette miliardi ed è stato detto che era poco. Posso dirlo? La storia dice che è stato poco rispetto a quello che è successo. E noi per i prossimi cinque anni mettiamo nove miliardi? Secondo me, ne occorrono il doppio (18), il triplo (27), il quadruplo (36, che è un numero non a caso, visto che è l'equivalente del MES). Io voglio un luogo nel quale poter dire che la sanità non va messa in secondo piano. Vi sembra normale che nel Next generation EU ci siano tre miliardi di euro turismo? Il turismo è la voce principale per la ripartenza, in particolar modo del Sud, e non solo. Ma vi sembra normale che il Parlamento stia zitto mentre la Germania della Merkel - che trascorre le vacanze in Italia, in Alto Adige o a Ischia

le dico con molta chiarezza che siamo pronti a discutere di tutto in un dibattito parlamentare aperto e franco. Non siamo disponibili a utilizzare la legge di bilancio come il veicolo nel quale si introduce quello che abbiamo letto sui giornali. In questo inserisco una vicenda altrettanto importante, relativa alla fondazione dei servizi segreti. servizi segreti. Se è vero, non possiamo immaginare di avere una fondazione a cui, al Copasir, le forze politiche, in modo pressoché unanime, dicono di no, mentre sui giornali leggiamo che verrà comunque inserita in legge di bilancio. Quindi, per giocare in maniera pulita e trasparente, se ci un provvedimento che tiene la *governance* del Next generation EU e un provvedimento che tiene la fondazione dei servizi segreti, noi votiamo contro. lo diciamo con molta lealtà; lo diciamo prima e invitiamo tutti a fermarsi finché si è in tempo. Quando, infatti, pensiamo ai servizi segreti, mi lasci dire che il 17 aprile 2015 un peschereccio italiano fu bloccato dai libici e portato via, ma nel giro di sei ore, l'allora Presidente del Consiglio chiamò l'allora autorità delegata e mandammo la Marina militare a riprendere quei quattro pescatori. Domani saranno centouno giorni che 18 pescatori sono nelle mani dei libici senza che nessuno muova un dito per questo. Signor Presidente, a chi dei suoi collaboratori continua a chiamare le redazioni dei giornali per dire che noi siamo alla ricerca di qualche poltrona comunico che, se ha bisogno di qualche poltrona, ce ne sono tre - due da Ministro e una da Sottosegretario - a sua disposizione in più. Se lei, invece, ha desiderio di ragionare sul serio e concretamente per il bene del Paese, spieghi ai suoi collaboratori che chiamano le redazioni che questo non è un *talk show* o il «Grande Fratello», perché questo è il Parlamento, questa è la politica e questo è il coraggio che Italia Viva ha e che spero abbiano altri.

intanto saluto il collega Renzi che usa le parole dell'opposizione. Ha strappato anche degli applausi da questa parte.

ha evitato accuratamente di approfondire la questione centrale, il nodo di fondo, ovvero la riforma del MES. Oggi noi siamo chiamati a un atto importante e suscettibile di gravità per la Nazione. Siamo chiamati, almeno formalmente, a dare un mandato al Governo sulla modifica del fondo salva Stati: questione che era stata accantonata, dopo essere stata affrontata con le note frizioni all'interno della vostra maggioranza, e discussa anche in Parlamento, il luogo deputato per farlo e dove è stata espressa contrarietà.

il ministro Gualtieri, nella riunione dell'Eurogruppo, in assenza di un mandato, ha dato il consenso italiano alla riforma e il MES è diventato, purtroppo, il fulcro nella gestione della crisi delle Nazioni dell'eurozona e questa è - a nostro avviso - la vergognosa ambizione della riforma. Della riforma del Meccanismo europeo se ne parla - l'abbiamo detto in molti - dal 2017, ma solo ora *hic et nunc* - guarda caso - diventa necessaria. Perché diventa un obbligo? E perché volete tanto una riforma che abbassa la soglia della maggioranza qualificata, che di fatto esclude - dal diritto di veto, conservato - guarda caso - da Francia e Germania, che detengono le quote maggiori all'interno del MES? Perché volete una riforma che trasferisce il potere decisionale in materia economica all'interno dell'organismo? E, soprattutto, perché legittimate il peggiore dei ricatti? Lo hanno ammesso apertamente esponenti della maggioranza dicendo che la riforma è pessima, ma serve. Insomma, si riprende quel *refrain* insopportabile e malato: "ce lo chiede l'Europa".

contro gli effetti della pandemia da Covid. La verità è che avete già deciso tutto non ora e non qui. Avete già deciso - come ricordava il collega Urso - che ricorrerete al MES sanitario e, infatti, nel *recovery plan* avete previsto per la sanità solo nove miliardi, di cui aggiungo - 4,2 per la ricerca e 4,8 per l'assistenza territoriale e la telemedicina. Sono decisamente un po' pochini in un Paese in piena pandemia, al quale avete promesso protocolli di cure domiciliari che non si sono invece mai visti, ma ne parleremo. Votando per la riforma del MES, imboccate definitivamente la strada che vi hanno indicato la Francia e la Germania e anche questo non da ora, ma dall'inizio di questo Esecutivo: una strada e un abbraccio mortale appunto, la modifica del MES e - Fratelli d'Italia lo sottolinea - la ristrutturazione del debito. Come stamane ha detto Giorgia Meloni intervenendo alla Camera, l'accesso al MES sanitario, con le sue condizionalità un aspetto che curiosamente non è stato modificato - è una delle tappe che ci porterà a un sostanziale commissariamento dell'Italia, con la ristrutturazione del debito, con con i prelievi forzosi dai conti correnti, con i nostri titoli di Stato a rischio, sui quali si può innescare una spirale speculativa e, ancora, con la polverizzazione dei nostri risparmi e magari anche con la patrimoniale. In sostanza, cari colleghi, si realizza il disegno tedesco dell'alto debito pubblico italiano ripagato con i risparmi degli italiani e, di fronte a questa evidenza, voi avete il coraggio di dirci che noi usiamo uno slogan quando gridiamo che il MES non serve all'Italia, ma che sono i soldi italiani che servono a garantire le banche francesi e tedesche piene zeppe di derivati. diciamolo: vi fa paura perché è la verità. Vedo che avete trovato un accordo all'interno della vostra maggioranza, dopo le finte minacce e le prove muscolari fatte a favore di telecamera; dopo le piroette stellari che hanno visto passare il MoVimento 5 Stelle dal dogma del No MES al mantra «Siamo responsabili, quindi sì alla riforma, anche se peggiorativa», per cui MES ni, anzi sì,

di deroghe che dovete giustificare al vostro elettorato. Ci lasciano attoniti le vostre giustificazioni alla capriola sul sì alla riforma del MES. Oltre al cedimento, che non vi fa onore, e alla legittimazione a quel ricatto di cui parlavo, mi voglio riferire anche alle dichiarazioni del ministro Di Maio che candidamente dice resta il no dei 5 Stelle al MES - non si sa dove resti - ma bisogna votare la riforma perché la posta in gioco è la sopravvivenza del Governo. - sarebbe quasi risibile in un altro contesto - un po' bambinesca, per la quale chiedete di votare la riforma, ribadendo però che tanto al MES noi non accederemo mai: altra grande bugia. Le vostre contraddizioni sono evidenti. Abbiamo tutti ascoltato anche adesso che cosa pensa il collega Renzi della *task force*,

dovrà decidere se fare retromarcia o cogliere la sfida finale e cruciale. Il centrodestra resta invece compatto

misure di sostegno per le filiere economiche più colpite dalla crisi e altresì di togliere - attenzione - quell'immunità concessa al MES e ai suoi dirigenti - immunità di cui non parlate mai mai - nonché le procedure di ristrutturazione del debito. Fratelli d'Italia voterà contro questa riforma, che rafforza il MES in qualità di super creditore e gli consente di sindacare su quali debiti siano o meno sostenibili dai tratta di un meccanismo che favorisce le consorterie europee, l'asse franco-tedesco e la linea di credito per i Paesi cosiddetti virtuosi, quelli che hanno il rigore nei conti pubblici, per capirci. Penso all'Olanda, che non è solo tulipani, ma è anche un paradiso fiscale che ogni anno toglie

verso quei Paesi che dissentono nei confronti del pensiero unico europeo. Cari colleghi, quando votate pensate che oggi ognuno di noi fa una scelta. Oggi questa maggioranza sceglie la strada dell'asservimento alle burocrazie europee, cede al ricatto e sacrifica gli interessi gli interessi dello Stato sovrano. Il nostro no a questa riforma è ontologico, è patriottico, è la difesa dell'Italia dalla dittatura economica del MES, è la difesa della sovranità nazionale dai *Diktat* europei. Se qualcuno mi ha insegnato che più buio che a mezzanotte non è, voi siete la mezzanotte della politica e state lasciando il popolo italiano - che lei non ha mai nominato nel suo discorso, signor Presidente, neanche una volta - nelle maglie strozzine dell'Europa, senza se e senza ma.

l'ONU ha richiamato tutti quanti noi e anche questa Aula, anche i Parlamenti, anche responsabilmente tutti i Governi del mondo,

quello che è accaduto a questo pianeta e al mondo, e le tante sofferenze che stiamo vivendo sono strettamente collegate alle crisi ambientali; noi le dobbiamo

impegna il Presidente del Consiglio e l'Europa a porre con forza il raggiungimento della neutralità climatica; a ridurre le emissioni di almeno il 55 per cento; ad agevolare un ulteriore obiettivo che forse l'Europa finalmente è in grado di darci. Questa è la nuova Europa, signor Questa è la nuova Europa, signor Presidente, che noi abbiamo voluto fortemente, anche quando era un'altra Europa; abbiamo combattuto per questo. Noi dovremmo essere orgogliosi

Questo sarà l'unico modo per poter far sì che nel nostro Paese, in Europa e a livello planetario si possa intraprendere la strada del progresso. Questo è il punto. L'occupazione, l'equità sociale si potranno raggiungere solo e unicamente se noi imboccheremo decisamente questa strada. È la questione più urgente all'attenzione del Consiglio europeo. Poi c'è il MES. Bene, abbiamo trovato

è un dibattito unico: siamo l'unico Paese europeo in cui si discute e ci si accapiglia sul MES; siamo l'unico Paese europeo in cui c'è il partito dei fondamentalisti del MES e il partito contro il MES.

e su questo dovremmo essere patrioti, visto che ho sentito usare questa parola. Infatti, se si vogliono fare fino in fondo gli interessi

riprendere il cammino degli ideali europei e degli ideali di integrazione europea. Questo significa oggi essere europeisti. Arriviamo a noi. abbiamo fatto varie volte scelte difficili e complicate; e arrivo al tema che adesso sta tanto appassionando i commenti:

chi più di noi ci tiene alla centralità del Parlamento? In quest'Aula noi abbiamo combattuto per far rispettare il Parlamento, anche contro le scelte che dal punto di vista costituzionale andavano dall'altra parte.

fare sintesi. *(Applausi)*. Lei è il Presidente del Consiglio e saprà fare sintesi. Noi siamo molto contenti

Nessuno più di noi - e lo dico a qualcun altro - è lontano dalla cultura dei commissari a cui si è fatto continuamente ricorso e dalla cultura della deroga.

*(PD)*. Signor Presidente, signor Presidente del Consiglio, membri del Governo, autorevoli colleghi, sono giornate difficili, complesse, che passano fra alti e bassi. bassi. Ho ascoltato gran parte del dibattito al Senato e anche una buona parte del dibattito alla Camera. Sono stato amareggiato nell'ascoltare, in particolare da esponenti di una parte dell'opposizione, termini molto pesanti, molto complicati da accettare nel momento che stiamo attraversando, anche considerando ciò che ci eravamo detti nel recente passato, parlando di collaborazione istituzionale, di unità di intenti, di richiamo al senso collettivo della comunità nazionale. Evidentemente così non è, tante bugie sono state dette. Ne prendiamo atto. Non è un bel momento, un bel passaggio, ma continuiamo a lavorare per il nostro Paese. Signor Presidente, intanto le dico grazie perché lei, il ministro Di Maio, il ministro Gualtieri e il ministro Amendola avete ricostruito la credibilità del nostro Paese in Europa vi dobbiamo ringraziare per questo. *(Applausi)*. Lo avete fatto con senso dello Stato e dell'interesse nazionale. Lo avete fatto mantenendo gli impegni che abbiamo preso,

nell'Europa il contesto nel quale ricrescere e ripartire dopo una crisi così difficile. La riforma del MES sta all'interno di questo percorso di serietà da parte nostra e di atti concreti verso il nostro Paese da parte dell'Europa. All'interno del provvedimento di riforma che lei andrà a sostenere - e noi siamo molto felici di questo - nelle prossime ore, sono comprese le scelte di politica ambientale come vera priorità per il futuro del nostro Paese, del nostro continente, del nostro Pianeta. Una massa di investimenti mai vista prima trasformeranno l'Italia e la nostra economia e ci permetteranno di ripartire.

Quindi sviluppo digitale, formazione e istruzione a tutti i livelli, come grande momento nel quale il Paese si dovrebbe ritrovare investendo nelle future generazioni. Poi ci sono i temi della politica estera: il Mediterraneo, la centralità dell'Italia, i rapporti con Paesi importanti come la Turchia, con il Nord Africa. Certamente anch'io mi associo all'appello sull'attivismo del Governo, affinché i nostri connazionali vengano presto liberati e abbiano la possibilità di trascorrere il Natale nelle loro famiglie *(Applausi)*, perché la situazione che stanno attraversando è inaccettabile. menziono la vicenda della Brexit. Io vivo come con grande disagio questi momenti, ma so che lei ci rappresenterà adeguatamente in quel contesto. Del resto, l'abbiamo detto fin dall'inizio, fin da quando questo Governo è nato sotto l'emblema dell'Europa: ci siamo trovati, insieme al MoVimento 5 Stelle e alle altre forze politiche, in Europa avendo una visione sull'Europa dei diritti e delle opportunità per le future generazioni; l'Europa del ritorno alla politica, al senso alto della politica; l'Europa dello sviluppo, del lavoro, della distribuzione della ricchezza creata tramite un'economia che cresce. Per questo i fondi di Next generation EU sono la grande sfida del futuro; una sfida che noi non possiamo mancare, in cui la *governance* che ci viene richiesta è uno dei passaggi centrali ed essenziali. Sono pragmatico, leggo i giornali e poi cerco di informarmi. In realtà aspetto, signor Presidente del Consiglio, che il Governo ci faccia arrivare presto una proposta. Io che credo, come molti di noi, nel Parlamento e nelle sue funzioni specifiche, so che il Governo ci invierà una proposta che noi avremo l'opportunità di esaminare, analizzare ed eventualmente anche di modificare con le indicazioni che i Gruppi parlamentari avranno l'opportunità di dare. Signor Presidente del Consiglio, su questo lei ce la deve mettere tutta: costanza, dialogo, confronto, coinvolgimento sulla *governance* così come sul piano. Allora permettetemi di ricordarlo: il Parlamento italiano, guardando in giro per l'Europa, è uno dei più coinvolti, e lo prendo a vanto della nostra azione nei confronti del Governo. Do atto in particolare al ministro Amendola di aver sempre posto su questo piano il confronto con il Parlamento; e così deve andare avanti. Lo ricordo a chi se lo fosse scordato: il 12 e 13 ottobre abbiamo avuto un confronto parlamentare, abbiamo votato degli atti di indirizzo precisi. noi pretendiamo dal Governo - ma il Governo credo che senz'altro lo farà - un passaggio intermedio di verifica per approvare il piano definitivo, perché questa è la funzione del Parlamento. Il Governo faccia il Governo e noi facciamo il Parlamento, fare sconti a nessuno, semplicemente nell'interesse del nostro Paese. Parlamentarizzare il confronto è stato un atto opportuno e necessario di coinvolgimento, e questo coinvolgimento, signor Presidente del Consiglio, lo dobbiamo allargare. Come Partito Democratico, chiediamo che sia il più ampio possibile nei confronti della società civile, delle imprese, dei sindacati, delle Regioni e degli enti locali. È ovvio che debba essere così, perché l'Italia del futuro dipende da questo e noi non possiamo fare nessun passo indietro. Ma non mi sembra che da parte del Governo ci sia questo desiderio. L'ho detto prima, forse anticipando - e sbagliando - in un comunicato pubblico. Mi aspettavo da lei un Consiglio dei ministri questa sera. Vorrei da lei presto un Consiglio dei ministri che non finisca fino a quando non ci sarà l'accordo da inviare al Parlamento. Poi starà noi fare la nostra parte, signor Presidente del Consiglio. Lei venga con una proposta e noi avremo la forza la determinazione di verificarla, di prenderla in considerazione fino in fondo e di rimandargliela con eventuali modifiche, se sarà necessario. Signor Presidente del Consiglio, concludo: a lei il mandato di continuare a rappresentarci, di continuare quell'azione di valorizzazione del nostro Paese, con contributi effettivi, indirizzati, che permettano all'Italia e all'Europa intera, insieme, di vivere i prossimi dieci anni come anni di cambiamento, di crescita, di sviluppo, di distribuzione della ricchezza.

Presidente del Consiglio, Ministri, Vice Ministri, Sottosegretari, colleghi, ho sentito dire molte cose che condivido, moltissime, anche da parti da cui non mi aspettavo di sentirle arrivare: dal padre putativo di questo Governo, che peraltro ha continuato a mantenere votando raffiche di fiducie che lo hanno stabilizzato. una punta di pentimento; noi avvocati diremmo «ravvedimento operoso ed attivo». Se questa punta di pentimento avrà un seguito è importante che noi tutti lo si sappia da subito perché credo che l'Italia sia veramente allo stremo e non ne possa più di questi teatrini. Signor Presidente del Consiglio, prendiamo molto sul serio il ruolo che lei domani avrà al Consiglio dell'Unione europea. L'ordine del giorno è importantissimo; lei dovrà rappresentare l'Italia e gli italiani e non dovrà dire in Europa - non lo farà, ne sono convinta

vede sicuramente, l'Italia che è stata descritta dall'ultimo rapporto Censis, che ha un sottotraccia spaventoso: la paura nera; gli italiani stretti in una morsa tra la paura della malattia e la paura della povertà la paura di non riuscire più a riappropriarsi della loro normalità: la loro vita normale, il loro lavoro, le loro famiglie, i loro dipendenti, il loro tutto che adesso è diventato niente. Signor Presidente, lei sicuramente vedrà quelle 350.000 aziende a rischio chiusura, quel milione di posti di lavoro perso a dicembre; lo vedrà e lo deve portare in Europa, e deve fare in modo che l'Europa sia in condizioni di aiutarci. Lei vedrà sicuramente 5,5 milioni di persone che sono scivolate in una povertà tale da rendere difficile mettere insieme il pranzo con la cena in un giorno; 8 milioni di persone che hanno denunciato un drastico, drammatico peggioramento della loro condizione economica e sociale. Il 66 per cento degli italiani dice

Un'Italia ferita dalle alluvioni, dalle montagne di fango con cui si sono svegliate porzioni d'Italia a cui portiamo tutta la nostra vicinanza, tutto il nostro affetto *(Applausi),* ma che devono essere supportate economicamente per dare la misura di quanto noi teniamo a loro. A proposito di tenere a loro, signor Presidente, ho sentito che il suo padre putativo lo ha ricordato: li vogliamo portare a casa quei 18 pescatori che da cento giorni sono prigionieri in Libia? *(Applausi).* La prego, approfittando della quarantena del Ministro degli affari esteri, li vogliamo riportare a casa? Signor Presidente del Consiglio, prendo molto sul serio quello che lei farà domani. Tutti noi lo stiamo prendendo molto sul serio. debba andare in Europa consapevole del fatto che per chiedere i soldi - gliel'ho già detto una volta - bisogna avere le condizioni per farlo. Bisogna avere le carte in regola, bisogna presentarsi con documenti

mettete tre miliardi sulla cultura e il turismo? *(Applausi)*. Tre miliardi sulla cultura e il turismo; 9 miliardi sulla sanità; ma lo vogliamo prendere questo MES sanitario? 37 miliardi a disposizione dal 1 giugno, che è altro rispetto alla riforma del Trattato del MES che non ci piace, perché pregiudica l'Italia. La vogliamo prendere quella linea di credito che possiamo spendere per gli ospedali, per i tamponi e per i vaccini? Per i vaccini di adesso, per i vaccini di poi, per le terapie intensive, per i polmoni d'acciaio; li vogliamo prendere? Basta pregiudizi ideologici. Se non si chiamasse MES, ma si chiamasse Ugo o Giuseppe li avremmo già presi e avremmo evitato ritardi ed errori di questo Governo. Signor Presidente del Consiglio, domani lei incontrerà i suoi omologhi. Chieda a loro se per caso hanno deciso a chi far gestire gli *action plan* del *recovery plan*, che peraltro sono già *on line* in Francia in Germania, con tanto di bandi e tempi di attuazione delle opere e dei servizi da settimane. se hanno intenzione di farli gestire dal Governo o da un esercito di nuovi burocrati a spese del contribuente, comandati da lei. Secondo me le risponderanno in coro «dal Governo», perché questa è la risposta giusta. Il Governo si deve assumere le sue responsabilità e visto che lei ha i Ministri più bravi del mondo, per quale motivo li vuole chiudere nello sgabuzzino delle scope, delegittimandoli e facendo lavorare un gruppo di esperti non meglio identificati? Un altro autorevole Ministro del suo Governo qui presente ha definito questa questa *task force* «struttura di missione»; non ricordo più com'è stata chiamata, ma l'ha definita «in odore di incostituzionalità». Sono d'accordo, anzi mi domando (se qualcuno lo sa mi risponda): dove sono finiti i professionisti dello sdegno democratico, i cantori della centralità del Parlamento, i moralisti in servizio permanente effettivo? #cimancate Ci mancate. Sono in sonno, come la bella addormentata, ma l'incantesimo finirà quando il centrodestra tornerà al Governo. Cerchiamo di farlo presto. Anzi, se il padre putativo fosse conseguente con quello che ha detto, potrebbe essere prestissimo. Signor Presidente del Consiglio, lei sa bene che in Europa bisogna contare, non compiacere. Stare in Europa non significa essere in prima fila per la *photo opportunity* o scambiarsi cortesie con i capi di Stato e di Governo. Significa difendere gli interessi del nostro Paese. Questo le chiediamo di fare, perché l'Europa è come un *club* inglese: ci si entra se si è soci; per ottenere le cose bisogna seguire le usanze della casa, ma bisogna imparare a usarle bene; non bisogna battere i pugni sul tavolo, ma non bisogna parlare a voce troppo tenue, sennò non ti sentono. Sono tutti amici, sì, ma anche molto competitivi tra di loro, perché vogliono tutti salire sulla poltrona più bella, vogliono tutti sedersi al posto migliore del tavolo e vogliono tutti prendere il premio più ambito. Allora, signor Presidente del Consiglio, bisogna farsi valere in Europa. Bisogna farsi sentire, bisogna che il suo *recovery plan* sia vero, condiviso. Ho sentito dire «condividiamolo con il Parlamento». Io riconosco al ministro Amendola professionalità e onestà intellettuale. Ministro Amendola, lei pensa veramente che quel rapido passaggio in Parlamento sia stato sufficiente per far sentire l'impronta l'impronta parlamentare su quello che è stato fatto fino ad ora? Ma ci sono le schede, ci sono le motivazioni, ci sono delle idee, oltre ai numeri a capocchia e a vaghi argomenti? Altrove ci sono rischiamo uno svantaggio competitivo terribile, rispetto a chi, in Europa, si sta già posizionando. Noi no e lo dobbiamo fare subito. Signor Presidente, vede, non c'è nessuna vena polemica in questo:

proposito della riforma del Trattato del MES, accettiamo di sottoporci a qualsiasi analisi del sangue di coerenza. È dal 2013 che diciamo che la riforma del Trattato del MES, così strutturata, non funziona, perché penalizza l'Italia, sottraendola dal pacchetto di mischia dei decisori delle decisioni importanti, e togliendo democrazia comunitaria all'azione del Trattato del MES, ci costringe a dare soldi quando non vogliamo e, visto che è sottoposta alle condizionalità del debito e del *deficit*, rischiamo di non avere soldi quando ne abbiamo bisogno (quei soldi che noi abbiamo conferito). Signor Presidente del Consiglio, entrando nel *club* inglese, deve promuovere il metodo solidale non il metodo intergovernativo, rigorista, lacrime e sangue, che piace tanto ad alcuni Paesi, che in questo momento stanno trattando l'Europa come un condominio, dove chi ha più millesimi decide per tutti. Non può funzionare così. signor Presidente del Consiglio, abbiamo capito che siete fragili e divisi, avete problemi interni, non riuscite a mettere giù le motivazioni dei vostri argomenti, perché non siete d'accordo su nulla, neanche su come stare seduti al tavolo europeo. Signor presidente Conte, lei in questo momento non rappresenta però solo la sua maggioranza, ma rappresenta gli italiani e un'Italia ferita, che ogni giorno, con sofferenza, sacrificio, coraggio e responsabilità affronta il Covid. Per loro deve lavorare *(Applausi)* e, come un direttore d'orchestra, deve dare le spalle al suo pubblico e inchinarsi agli italiani, non all'Europa. Su questo, signor Presidente, per la difesa di tutti quelli che stanno affrontando il dolore e la sofferenza - 60.000 morti, amici: è un prezzo spaventoso! prezzo spaventoso! - per tutti quelli che stanno soffrendo ora e per tutti quelli che non ci sono più, noi ci saremo, per tutelare i loro diritti, sempre. Noi di Forza Italia, noi del centrodestra, in ogni luogo, nell'Europarlamento, in Parlamento, nelle piazze e nel Paese, in ogni modo possibile e, come direbbe qualcuno, *whatever it takes*, noi ci saremo.

dedicherò solo due brevi passaggi a due motivi di critica su quello che abbiamo ascoltato e il resto lo dedicherò all'idea di Italia che secondo me tutti dobbiamo avere in testa, lasciando proposte su cui avremmo voglia di confrontarci. Sta poi a voi, colleghi, scegliere se è il momento del litigio, del rimpasto, della divisione, della confusione, dei documenti di 17 pagine o se pure è venuto il momento di guardarsi negli occhi, rendersi conto del fatto che abbiamo 60 milioni di persone dietro di noi ed essere responsabilmente conseguenti. Potremmo percorrere una via più semplice: rappresento un movimento che da due anni e mezzo è il primo partito del Paese, col 25 per cento dei consensi. Facciamo parte di una coalizione - non dico «rappresento», perché non voglio urtare la suscettibilità di nessuno - e il centrodestra era, è e rimarrà maggioranza politica, economica e sociale del Paese. Quindi, con una scelta egoistica, potrei dire: assistiamo al fatto che voi continuate a commettere degli errori, ci limitiamo a denunciare gli errori che state commettendo e aspettiamo, prima o poi, di arrivare al voto - perché, prima o poi, al voto si arriverà dicendo che avete fatto il male del nostro Paese e che adesso tocca a noi. Non vorrei però che fossero tutti gli italiani a pagare gli errori che qualcuno sta commettendo. *(Applausi)*. Quindi con tutti i nostri limiti vorremmo segnalare quello che a nostro modesto avviso non va, per provare a porvi rimedio insieme *(Applausi)*. Sui temi europei vorrei dare due spunti al volo, senza ripetere quello che già in tanti hanno detto. Si parla giustamente anche in quest'Aula di diritti umani; è sacrosanto,

da fuori che dal 2000 ad oggi i contribuenti italiani ed europei hanno dato alla Turchia 50 miliardi di euro, che l'anno prossimo è previsto un altro miliardo di euro a quello che è un regime islamico che incarcera avvocati, giornalisti e oppositori. Io sono stufo di finanziare un regime islamico che non conosce il significato della parola democrazia. La invito quindi a portare a Bruxelles questa voce forte; mi dicono però che il presidente Conte non può alzare troppo la voce nei confronti della Turchia perché ci ricatta sul tema dell'immigrazione ai confini Est e ai confini Sud; basta con il ricatto nel nome dell'immigrazione clandestina; difendiamo i confini di questo amato Continente. *(Applausi)*. Difendiamo i confini italiani ed europei, invece di pagare chi fa il lavoro sporco. Mi auguro che abbia il coraggio di portare questa voce di libertà e di diritti umani. Il MES, come abbiamo già detto, dal nostro punto di vista è un Robin Hood al contrario, che porta via soldi a chi ne ha bisogno per salvare le banche dei tedeschi che non ne hanno bisogno. Se io dovessi riassumere, l'idea è questa, con l'obiettivo finale di dire che l'Italia ha bisogno di quei soldi, ma prima di accedervi deve fare altri tagli, come abbiamo già fatto in passato, chiudendo altri ospedali e altre caserme dei Vigili del fuoco. No. Errare è umano, perseverare sarebbe diabolico. *(Applausi)*. Stiamo morendo di austerità, basta con i tagli e le chiusure. proposte, io penso che l'intero centrodestra sia disponibile non da dopodomani, ma da domani a confrontarsi con lei e coi suoi Ministri su alcuni temi molto concreti.

ma importante dal mio punto di vista, che io invito il Governo a tenere in debita considerazione, perché se tutte le Regioni sostengono la stessa cosa non è una guerra dei sovranisti contro questo Governo, ma una proposta che probabilmente ha senso. L'Italia è la capitale mondiale del volontariato; ora qualche burocrate - sicuramente lei non ne è a conoscenza - ha inserito negli ultimi provvedimenti una norma che obbliga tutte le associazioni di volontariato italiano, anche le più piccole, ad aprire una partita IVA e a emettere fattura. È una follia che non sta né in cielo né in terra. *(Applausi)*. Lasciamo che il mondo del volontariato occupi il suo tempo facendo volontariato, non compilando moduli per poi chiedere l'esenzione IVA. Passando

cento venga destinato a progetti di abbattimento delle barriere architettoniche: lo 0,1 Penso sia giusto che questo Parlamento all'unanimità dia una risposta immediata a questi sei milioni di cittadini italiani, che non sono cittadini di serie B. vi invito ad ascoltare con più attenzione le richieste dei sindacati; da parte mia è una richiesta che può sembrare abbastanza strana, ma è un momento in cui non bisogna chiudersi in recinti ideologici. Parlare di infermieri eroi e poi non concedere neanche un euro di aumento agli infermieri e al personale sanitario è una presa in giro che queste lavoratrici e salute al capitolo lavoro, gli italiani in questo momento non sono preoccupati per il rimpasto evocato da Renzi, temuto da Zingaretti, deprecato da Mattarella, che vedo molto attivo con dei retroscena sui giornali e mi auguro che sia altrettanto operativo e attento nel difendere le prerogative del Parlamento, che rappresenta la democrazia e l'unità di questo Paese. *(Applausi)*. Ci sono a fine anno milioni di lavoratori autonomi non tutelati che hanno fatturato zero e dovranno versare i loro minimi alle casse di previdenza. Il problema non è il contributo alla cassa forense dell'avvocato Conte, che non ha problemi, il problema riguarda quegli agenti di commercio, quegli architetti, quei geometri, quegli avvocati e quelle partite IVA che non hanno incassato una lira e non possono pagare migliaia di euro alle loro casse previdenziali. *(Applausi)*. Spero che questo sia argomento di dibattito unitario. Ci sono alcune aziende strategiche per il Paese, penso a due in particolare che meriterebbero più attenzione. L'Ilva; è folle che in un momento in cui mezzo mondo avrà bisogno di acciaio per essere ricostruito, noi rischiamo di svendere al primo miglior offerente un patrimonio che non è solo tarantino, ma è un patrimonio italiano, che è quello delle Acciaierie di Taranto. Difendiamo l'Ilva e la produzione di acciaio italiana

che gridano giustamente «onestà, onestà» di non mettere a rischio un'azienda strategica per il patrimonio italiano e di mettere in sicurezza un'azienda che rischia di essere scalata e acquistata sottocosto dal primo investitore che arriva dall'altra parte del mondo. Non regaliamo l'acciaio e la difesa magari ad un investitore cinese che è pronto ad arrivare domani mattina con i contanti nella borsa. *(Applausi)*. Noi siamo disponibili a lavorare sul tavolo del rilancio dell'Ilva. Se nei fondi del *recovery fund* ci fosse anche il ponte sullo Stretto di Messina, uniremmo due necessità in una sola. Daremmo un'infrastruttura attesa da decenni a una parte d'Italia che è isolata e daremmo commesse per decenni a un'azienda che altrimenti rischia di essere svenduta. Inseriamo allora questo benedetto ponte sullo Stretto di Messina nel futuro che unisce il Paese da Nord a Sud. Due temi finali che mi stanno particolarmente a cuore. Il primo è la scuola;

avrò detto cinque volte in quest'Aula, se lei e il ministro Azzolina riteneste, noi domani come centrodestra saremmo al tavolo di confronto perché dire il 7 gennaio riaprono indistintamente le scuole, significa mettere a rischio la salute di milioni di studenti, di milioni di familiari degli studenti e di un milione di insegnanti. *(Applausi).* Se nel frattempo non si è fatto nulla sul trasporto pubblico locale, sull'areazione delle classi, sulla stabilizzazione degli insegnanti precari, dire oggi che il 7 gennaio rimanderemo a scuola tutti i nostri figli, rischia di essere una catastrofe. Parliamone prima per evitare di accorgerci dopo del danno fatto. Un'ultima riflessione sul Natale. Abbiamo parlato di Europa. Cosa fanno in tutti gli altri Paesi europei per limitare i contagi il il giorno di Natale senza dividere le famiglie e i cittadini? In Portogallo non c'è alcuna limitazione; in Francia non c'è alcuna limitazione.

in casa e non più di tre famiglie diverse. Giusto, non c'è alcun senso, alcuna giustificazione scientifica al fatto che solo in Italia si dica alla gente che il giorno di Natale non si può uscire dal recinto e dalla gabbia del proprio Comune. Signor Presidente del Consiglio, si metta la mano sul cuore e pensi a quei milioni di italiani soli, di donne e di uomini che almeno il giorno di Natale hanno diritto a un po' di affetto, a un sorriso. Penso ai genitori separati, al volontariato,

che metta insieme la tutela della salute con il diritto all'affetto; 6.000 Comuni italiani su 8.000 hanno meno di 5.000 abitanti; 1.500 Comuni italiani su 8.000 hanno meno di 1.000 abitanti: diritto alla salute sì,

la Lega e l'intero centrodestra sono a disposizione. Viva l'Italia delle libertà e dei piccoli Comuni!

stiamo attraversando giorni terribili e momenti difficili. Gli italiani hanno mostrato senz'altro di comprendere bene la necessità di certi sacrifici. Anzi,

l'impossibilità per quest'Assemblea di dibattere di temi che sono il futuro di questo Paese. Si tratta di temi europei: lo Stato di diritto, l'integrazione, la sicurezza, il Covid e i vaccini sono tutti temi che tracciano il futuro di questo Paese. In questa sede abbiamo invece sentito parlare di tutto e di più:

della quale abbiamo sempre detto: ti prego, prima della fine dell'anno vieni una volta e dacci una soluzione. Non replico a chi viene qua e porta il proprio volantino elettorale. La campagna elettorale ci sarà, ma questo non è il momento di venire in Aula e portare ciascuno il proprio volantino elettorale. Replico all'amico Matteo Renzi,

con frasi del tipo «lo dico per il bene del Paese» o «lo dico per il bene degli italiani». Non riusciamo a compiere un dibattito sull'Europa senza scivolare nella palude delle guerre tra bande e delle beghe di potere. Comprendiamo che all'orizzonte c'è una montagna di miliardi e questo stuzzica gli appetiti di tutti e qualcuno probabilmente si sente tagliato fuori. Noi questo lo comprendiamo, ma ciò che non capiamo e non giustifichiamo è che in tutto questo dibattito non ci sia stato un solo pensiero per le centinaia di cadaveri che ogni giorno stanno uscendo dai nostri ospedali,

per colpa di una malattia e di un'emergenza sanitaria che in questa Aula ancora viene utilizzata come un'arma politica. Lidia Menapace, che abbiamo commemorato questo pomeriggio, la patriota che ci ha lasciato lunedì, anch'essa per Covid-19, diceva che dobbiamo fare in modo che il luogo in cui viviamo sia il più umano possibile

un'Europa più umana, equa e solida. Oggi sappiamo che la nuova Europa passerà attraverso l'emissione di eurobond,

i temi banditi da Bruxelles sui quali il MoVimento 5 Stelle aveva scommesso già da quando si era deciso di diventare decisivi per la nomina della signora von der Leyen. Qualcuno ha detto che il MoVimento 5 Stelle ha compiuto una piroetta e, a un certo punto, è diventata europeista. No, è diventata europeista. No, noi siamo sempre stati fortemente eurocritici; noi addirittura diffidiamo ancora oggi degli europeisti della prima ora, di quelli che sostenevano la politica che andava a Bruxelles con il cappello in mano e tornava in Italia a fare macelleria sociale. Noi continuiamo ancora oggi a difendere e a sostenere i valori di solidarietà e contrastiamo quelli che allora hanno appoggiato la politica dell'*austerity*, la politica della finanza e delle banche.

Fate continuare. Avete parlato tutti e c'è stata attenzione su quanto hanno detto tutti. Fate parlare il senatore Licheri. e senatori, la risoluzione archivia definitivamente quella stagione. Vi invito a leggere la risoluzione non a far svolazzare cartelli o giornali. Leggete la risoluzione; leggete l'ultimo capoverso di pagina 13. Votiamo tutti questa risoluzione. Il Parlamento italiano sarà il primo in Europa a dichiarare ufficialmente che non vogliamo più alcun organo intergovernativo in Europa. Il primo Parlamento in Europa che certifica la morte anticipata del MES. Il primo Parlamento che dichiara superata la logica intergovernativa e terminata la filosofia del controllo del debito piuttosto che del sostegno al debito. Votiamo questa proposta di risoluzione. Il Parlamento italiano a pagina 13, nell'ultimo capoverso, dice testualmente: pretendiamo come cittadini italiani, ancora prima che parlamentari, una profonda riforma del Patto di stabilità e crescita prima della sua reintroduzione. Pretendiamo! Senatore Monti, con il dovuto e pieno rispetto, in questa proposta è scritto ciò che molti in passato non hanno avuto il coraggio di pronunciare: l'Italia è tornata protagonista nei tavoli delle grandi decisioni e non possiamo rischiare di gettare alle ortiche quel patrimonio di credibilità internazionale che ha acquisito il nostro *Premier*. Da poche ore un'agenzia *on line* indica Giuseppe Conte come il politico più influente in Europa in questo momento. *(Applausi).* È possibile che fuori siano diventati così? Allora usiamo il Covid come un acceleratore dei processi di cambiamento, pensiamo alla *green rule*, allo scorporo dal *deficit* degli investimenti sostenibili, al superamento delle regole di ingaggio della BCE e del *capital key*, alla radicale e profonda riforma del Patto di stabilità e crescita, che è il basamento sopra il quale è stata costruita la casa del MES. Altro che MES! Mi sto accingendo alla conclusione. Nessun Paese europeo vuole i prestiti del MES; in nessun Paese europeo si discute... Presidente, per cortesia.

Abbandoniamo questo dibattito sterile del MES. Nessun Paese europeo vuole i prestiti del MES e fin quando il MoVimento 5 Stelle siederà su questi banchi l'Italia non li prenderà mai, non li accetterà

...solo i cretini. Stiamo affrontando una pandemia terribile; milioni di persone sono in gravi difficoltà. Stanno per arrivare i miliardi del *recovery fund* e qualcuno parla di crisi di Governo? Oppure qualcuno parla di crisi di Governo perché stanno per arrivare i miliardi del *recovery fund*?

tutti uniti, siamo ancora più uniti di prima, perché siamo tutti dentro un sogno, quello di cambiare un'Europa dove le vecchie ricette non hanno funzionato. Se c'è la crisi di Governo, si riapriranno le urne. Noi non abbiamo paura delle urne, noi non abbiamo paura delle sconfitte. *(Commenti)*. PRESIDENTE. Per cortesia, fate concludere. Avete sforato tutti. Prego. Noi non abbiamo paura delle urne. Noi non abbiamo paura delle sconfitte, perché sulle sconfitte abbiamo fondato le nostre vittorie. Peccato solo che, alla fine, a pagare questo conto salato saranno sempre e solo i cittadini.

il Meccanismo europeo di stabilità costituisce la parte peggiore dell'Unione europea e rappresenta tutto ciò contro cui il MoVimento 5 Stelle si batte. Io vorrei ascoltare. Per cortesia, che ognuno stia al suo posto. Prego, senatore Crucioli. Esso incarna il primato della finanza sull'uomo ed è lo strumento per garantire che i crediti vengano ripagati anche a costo del sacrificio di interi popoli. È il randello contro gli Stati che restano indietro, lo strumento per sottrarre loro sovranità, a danno dei più deboli. È il regno dei verbali segreti e dell'immunità da qualsiasi giurisdizione. Avremmo dunque dovuto dare mandato al Presidente del Consiglio per chiederne una profonda riforma o per ingabbiare tale mostro all'interno di altri strumenti che ne mitigassero la nocività. Questa era la famosa logica di pacchetto. Invece stiamo mandando il Presidente a rinnovare l'adesione dell'Italia a questo trattato, autorizzandolo, anzi, ad approvare alcune riforme peggiorative. Il fatto che nella risoluzione si chieda che il Presidente si faccia promotore della modifica del patto di stabilità, della revisione del MES stesso e del raggiungimento di un accordo sullo strumento chiamato EDIS (*European deposit insurance scheme*) risulta contraddittorio. Come possiamo, infatti, conciliare tali richieste con l'ok al rafforzamento del MES che stiamo autorizzando? Il patto di stabilità che chiediamo di rivedere è il presupposto stesso dell'esistenza del trattato sul MES, che con il voto di oggi si vuole confermare e peggiorare. Non vi rendete conto, inoltre, che chiedere la modifica radicale del MES nello stesso documento con cui ne ribadiamo l'adesione risulta paradossale? Anche quanto affermato dal Presidente del Consiglio su tale punto mi pare non condivisibile. Se si vuole davvero riconsiderare in maniera radicale struttura e funzione del MES come lei ci ha detto, Presidente - non si deve andare in Europa e dare l'adesione ad una riforma che ne conferma e rafforza l'impianto. Quanto ad EDIS, tale strumento avrebbe dovuto essere approvato contestualmente alla riforma del MES, non prima il MES e poi forse EDIS. In conclusione, io temo che oggi il Parlamento stia armando inconsapevolmente la mano che domani potrebbe colpirci. La vostra visione delle magnifiche e progressive sorti dell'Unione europea è frutto di un errore prospettico. Io credo che l'urgenza di ribadire e rafforzare il MES non sia affatto un passaggio di un più ampio progetto di solidarietà europea, bensì la volontà di ribadire che la stagione degli aiuti per la pandemia...

che la stagione degli aiuti per la pandemia è temporanea e legata esclusivamente alla necessità che il nostro naufragio non trascini con sé l'intera situazione europea. Il bazooka della BCE non sparerà ancora a lungo: passata l'emergenza sanitaria ci verrà chiesto il conto e il MES è lo strumento. Oggi tutti noi ci esponiamo giudizio della storia: resti agli atti che ho lottato lealmente, con tutte le mie forze e fino all'ultimo contro questa risoluzione.

quando ero al liceo mi sentivo un po' stupido a dover spiegare il paradosso di Zenone secondo il quale, in una gara, Achille non avrebbe mai raggiunto la tartaruga alla quale aveva concesso un vantaggio iniziale. Oggi, però, vedo che c'è qualcuno più paradossale di Zenone, quasi uno Zalone. Ecco, Conte Zalone vorrebbe farci credere che la riforma del MES va votata ma non va attuata perché brutta, sporca e cattiva. Il paradosso che proponete è illogico, è un non senso, tanto quanto la tartaruga che sarebbe sempre più avanti rispetto ad Achille. Il MES lo prenderete. Sarete costretti a prenderlo perché ve lo ordinerà quella Bruxelles della von der Leyen che vi ha già obbligati alla riforma stessa. Quella Bruxelles da dove siete andati a prendere il ministro Gualtieri. La BCE non continuerà a lungo ad agire come se fosse un prestatore di ultima istanza, a comprare titoli sui mercati secondari, ad allargare le maglie del *capital key rule* o a forzare il suo ruolo sui tassi di interesse perché il libretto di istruzioni della BCE non prevede questo. Il Governo giapponese ha approvato ieri un altro piano di stimolo pari a 580 miliardi di euro. Così, quando la BCE smetterà di fingersi *market maker* i tassi di interesse si alzeranno e si giocherà alle regole dei mercati finanziari e siccome nessuno coprirà più le nostre spalle, ecco che il Governo dovrà accedere alla linea di credito del MES, altro che smantellarlo. Conte e Gualtieri promisero alla signora Ursula che saremmo stati disciplinati scolaretti e che l'Italia sarà pronta a ristrutturare il debito pubblico come vogliono i falchi, quindi imponendo ancora sacrifici, tagli e austerità. State tradendo il senso del voto delle ultime politiche: la maggioranza degli italiani voleva uscire dal sistema, dalla gabbia e per questo aveva premiato democraticamente le forze che si presentavano come antisistema. State completando la transizione dal popolo sovrano ai mercati sovrani, dai cittadini alle *lobby* sovrane e ai grembiulini sovrani. Avete svuotato questa Assemblea, non avete più pudore. Per reggere questo Governo di "euroinomani" il MoVimento 5 Stelle sta tradendo il programma che ha presentato agli elettori, sta tradendo i cittadini che volevano vederlo battagliare per difendere il popolo sovrano e chi combatte le giuste battaglie può morire, vero, e chi fugge, come state facendo voi, resterà vivo, almeno fino alla fine della legislatura. Ma tra molti anni a partire da adesso, siete sicuri che non sognerete di barattare tutti i giorni che avrete vissuto a partire da oggi per avere un'altra occasione, solo un'altra occasione per difendere la libertà degli italiani, per respingere il ricatto della finanza, per urlare che le regole di Bruxelles sono un ricatto infame? Voi dicendo sì oggi, state dicendo sì al MES. State omaggiando Caronte di un altro colpo di remo per spingere gli italiani verso l'euroinferno. No MES. Viva Italexit!

Signor Presidente, signor Presidente del Consiglio, colleghi senatori, credo che tra le tante critiche possibili al Presidente del Consiglio dei ministri, l'avvocato Giuseppe Conte, la più pertinente, e anche la più grave, sia quella di aver incartato se stesso e la nazione in una narrazione non vera. Abbiamo sentito elevare l'Italia a modello per la capacità di contenere il virus. Lo abbiamo sentito parlare di vigorosa ripresa dell'economia. Questo evidentemente non è vero. È grave che un capo di Governo forzi la realtà e ancor più grave che la forzi su un terreno così drammatico per la Nazione, la crisi sanitaria ed economica. Credo che chi si accinge a ricoprire funzioni di Governo e chi aspira a rappresentare un'alternativa credibile di Governo, debba evitare il rischio di cadere in errori simili, di forzare la realtà, sia pur non avendo le medesime responsabilità, e sia pure su terreni ben meno scivolosi ma non meno simbolici. Il realismo, credo, dovrebbe essere la nostra principale bussola e credo che la realtà sia che se noi del centrodestra, perimetro all'interno del quale sono stato solo e sempre rimarrò, fossimo al Governo, la riforma del MES l'avremmo approvata. E l'avremmo approvata come l'hanno approvata tutti gli altri Governi dell'eurozona; impegnandoci e impegnando la nostra capacità politica per temperarne nel tempo le storture e le criticità, che ci sono; ma l'avremmo approvata. L'avremmo approvata perché mai come oggi abbiamo bisogno dell'Europa, e mai come oggi l'Europa ha cambiato segno e senso: siamo passati - e non era facile immaginarlo - dalla logica intergovernativa alla logica comunitaria. E se non approvassimo quella riforma, metteremmo Noi avremmo approvato la riforma del MES perché è comunque meglio del MES originario, e se non passasse tale riforma ci troveremmo con il MES delle origini. L'avremmo approvata credo anche perché ce lo chiedono la Confindustria, il sistema bancario e le associazioni datoriali. L'avremmo approvata anche perché, diversamente, ci saremmo attirati quell'effetto stigma che, a torto, si ritiene che l'Italia si attirerebbe se accedesse al MES pandemico. Colleghi, viviamo tempi difficili e problemi complessi. Banalizzare la complessità dei problemi credo che pregiudichi la possibilità di risolverli, quando se ne avrà la responsabilità. Per queste ragioni, ringraziando i colleghi del Gruppo Forza Italia e il Capogruppo per il per il rispetto e la sensibilità dimostrata nel riconoscere le mie ragioni, non potendo naturalmente votare a favore della proposta di risoluzione del Governo, perché questo correrebbe il rischio di rendermi responsabile della sopravvivenza di un Governo che ritengo esiziale esiziale per il presente e per il futuro del Paese, non perché sia un Governo malvagio, ma perché è un Governo nato in stallo e che in stallo è rimasto, annuncio che non parteciperò al voto.

Signor Presidente, signor Presidente del Consiglio, membri del Governo, colleghi, a marzo 2018 il 33 per cento degli italiani ha dato fiducia ad un partito che si è presentato in Parlamento per smantellare il MES, punto di programma fatto votare ai cittadini iscritti alla piattaforma. Oggi, i cosiddetti portavoce faranno l'esatto contrario: non solo non smantelleranno il MES, ma addirittura daranno il via libera a una sua versione rafforzata. Diventerà così possibile, per una maggioranza semplice di detentori del nostro debito pubblico, chiederne la ristrutturazione, come ha voluto l'asse franco-tedesco fin dal vertice di Meseberg del giugno 2018. La Commissione europea non avrà più un ruolo paritario con il MES nella gestione dell'emergenza finanziaria dell'eurozona, la quale resterà in mano al solo MES, i cui membri oggi hanno ogni tipo di immunità e le cui sedi sono inviolabili. Con il Fondo di risoluzione unico i nostri contribuenti saranno chiamati al salvataggio delle banche altrui ed ogni tipo di erogazione di aiuti sarà subordinata alla valutazione di sostenibilità del debito, monitorata ogni sei mesi con condizioni sempre rivedibili. Lo dico soprattutto a voi che, nel tentativo di mantenere quel poco di sostegno elettorale che vi resta, non vi fate scrupolo di affermare che state solo dando il via libera alla riforma peggiorativa, ma che non ne chiedete l'attivazione. Troppo comodo. La verità è che lasciate la porta aperta a chiunque la vorrà attivare. Invece questa cosa andava fermata proprio adesso, come promesso agli elettori. Tutto questo

Prima di passare alle votazioni, avverto che, in linea con una prassi consolidata, le proposte di risoluzione

Comunico che è stato trasmesso dalla Camera dei deputati il seguente disegno di legge: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-*bis*, 391-*bis*, 391-*ter* e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del web e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale»